L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

il Documento di economia e finanza 2016, in linea con le previsioni di legge, illustra l'andamento macroeconomico del Paese, traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche e definisce gli indirizzi, sul versante delle politiche pubbliche, per il rispetto del Patto di stabilità e crescita europeo. Enuncia poi le modalità e la tempistica attraverso le quali l'Italia intende conseguire il consolidamento strutturale dei conti pubblici e perseguire gli obiettivi in materia di crescita, occupazione, innovazione, istruzione, integrazione sociale, energia e sostenibilità ambientale definiti nell'ambito dell'Unione europea.

In particolare, la prima sezione del Documento espone lo schema del Programma di stabilità, che contiene tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea dal nuovo codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi di politica economica da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. Nella seconda sezione sono indicate le regole generali sull'evoluzione della spesa delle amministrazioni pubbliche, in linea con l'esigenza, evidenziata in sede europea, di individuare forme efficaci di controllo dell'andamento della spesa pubblica. La terza sezione reca, infine, lo schema del Programma nazionale di riforma (PNR) che, in coerenza con il Programma di stabilità, definisce gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delineati dalla nuova Strategia Europa 2020. In allegato al Documento sono riportate una serie d'informazioni supplementari contenute in apposite appendici. il DEF 2016 evidenzia una situazione macroeconomica e di finanza pubblica tendenzialmente positiva sia con riguardo alle prospettive di crescita del nostro sistema economico che con riguardo all'andamento delle finanze pubbliche, pur non nascondendo le difficoltà emergenti dal contesto internazionale.

che si incrementa negli anni successivi, per effetto delle politiche del Governo, dell'1,4 per cento nel 2017, dell'1,5 nel 2018, e del 1,4 per cento nel 2019. Tale andamento influirà positivamente anche sul mercato del lavoro e il tasso di disoccupazione è previsto scendere fino al 10,6 Gli occupati e il monte ore lavorate aumenterebbero in tutto il periodo di riferimento e la maggiore produttività, accompagnata da una moderata crescita salariale, si rifletterebbe in una dinamica ancora contenuta del costo unitario del lavoro. Per quanto riguarda i contributi alla crescita del PIL, il Governo, per l'anno in corso e per quelli successivi, prevede una buona ripresa della domanda interna che, stante l'andamento di scorte ed *export*, da sola dovrebbe garantire il *trend* di crescita alla nostra economia ad un livello medio dell'1,4 per cento (ovviamente considerando la costanza delle esportazioni). Il dato che emerge è complessivamente positivo, soprattutto se paragonato con la situazione emergenziale degli scorsi anni per quanto riguarda gli andamenti della finanza pubblica, e mostra per il periodo di riferimento un andamento decrescente del *deficit* e della spesa per interessi ed un'incoraggiante crescita dell'avanzo primario, a dimostrazione che le misure di stabilizzazione dei conti pubblici iniziano a produrre i risultati attesi. Nel nuovo scenario programmatico il Governo prevede che l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche si riduca dal 2,3 per cento del 2016 all'1,8 per cento del PIL nel 2017 e allo 0,9 per cento nel 2018, portando quindi il saldo in lieve *surplus* nel 2019 (0,1 per Fra i dati maggiormente significativi si segnala l'andamento dell'indebitamento strutturale, che, sebbene in peggioramento nel 2016 rispetto alle previsioni del precedente DEF (0,7 punti percentuali rispetto al 2015),

assicurerebbe sostanzialmente il conseguimento dell'Obiettivo di medio termine (MTO) dell'Italia nel 2019, anno in cui il saldo è previsto al -0,2 per cento. La deviazione temporanea dal percorso di avvicinamento verso l'Obiettivo di medio termine rispetto alle precedenti previsioni è pertanto riconducibile all'esigenza di procedere speditamente, con una strategia organica, all'implementazione degli interventi per la crescita, in grado di incidere nel medio periodo sul potenziale di crescita del PIL e di migliorare la sostenibilità delle finanze pubbliche. Per queste ragioni, il Governo ha predisposto una Relazione al Parlamento, che verrà sottoposta all'autorizzazione parlamentare. La Relazione, come già accennato in apertura, contiene l'aggiornamento dei nuovi obiettivi programmatici di finanza pubblica, l'indicazione della durata e la misura dello scostamento, nonché il relativo piano di rientro, tenuto conto della durata e della gravità degli eventi da fronteggiare, fissando un sentiero di riduzione dell'indebitamento netto più graduale rispetto a quello programmato nella Nota di aggiornamento 2015, che assicura comunque il sostanziale raggiungimento dell'obiettivo di medio termine nel 2019. Fra gli altri dati positivi di finanza pubblica si sottolineano quelli relativi all'andamento del saldo primario e della spesa per interessi, che confermano il percorso virtuoso intrapreso verso il risanamento delle finanze pubbliche. del rapporto debito-PIL, infine, dopo una ulteriore crescita nel 2015 fino al 132,7 per cento del PIL, dal 2016 si avvia la fase di discesa, con una prima riduzione di 0,3 punti percentuali rispetto all'anno precedente, fino a raggiungere il livello del 123,8 per cento nell'anno terminale del periodo di previsione, con una riduzione complessiva nel periodo medesimo di circa 9 punti percentuali. seconda sezione del DEF sono riportate, fra le altre, le previsioni tendenziali dei conti economici delle pubbliche amministrazioni. Le entrate totali delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL presentano un percorso di diminuzione, passando dal 47,9 per cento registrato nel 2015

netto degli interessi in rapporto al PIL, dopo gli aumenti registrati negli anni 2013, 2014 e 2015, sono previste ridursi costantemente sull'orizzonte previsivo, fino a raggiungere il 39,9 per cento del PIL nel 2019.

La riduzione della spesa in conto capitale fra il 2015 e il 2019 è pari a -0,8 punti percentuali del PIL ed è comunque più contenuta di quella prevista per le spese correnti al netto degli interessi; processo destinato a continuare nel prosieguo del percorso di risanamento dei conti pubblici, al fine di creare una situazione della finanza pubblica in grado di supportare al meglio lo sviluppo e la crescita economica. Il fabbisogno del settore pubblico risulta in costante miglioramento fino a raggiungere, nel 2019, il valore positivo di 652 milioni di euro. Le stime per il 2016 indicano un fabbisogno del settore pubblico pari a Il Programma nazionale di riforma contenuto nella terza sezione del DEF definisce, in coerenza con il Programma di stabilità, gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità così come delineati e concordati in sede europea. Anche in relazione alle raccomandazioni dell'Unione europea di luglio 2015 il PNR compie una ricognizione delle misure adottate ed *in itinere*, nonché dei nuovi interventi che il Governo intende effettuare. Gli ambiti principali d'interesse del PNR concernono in particolare la competitività e gli investimenti per la crescita, con importanti misure per esempio per quanto riguarda l'utilizzo di fondi strutturali nel Mezzogiorno con il *masterplan*, le riforme istituzionali, la pubblica amministrazione e le semplificazioni, il mercato del lavoro e le politiche sociali, la riforma della giustizia, il sistema bancario e la finanza per la crescita, le privatizzazioni, le politiche per la concorrenza, l'istruzione e ricerca, la rimozione degli squilibri territoriali, la lotta alla povertà, l'imposizione fiscale e la riforma della legge di bilancio. Il DEF 2016 illustra pertanto i principali obiettivi di politica economica ritenuti necessari per accompagnare il suddetto processo di crescita. Fra questi, si evidenziano gli interventi prefigurati nel DEF volti a sostenere la ripresa economica, la riduzione del prelievo fiscale, le misure per convogliare il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo su un percorso di riduzione, agendo soprattutto sul denominatore dello stesso rapporto, cioè la crescita, e consolidando così la fiducia dei mercati per favorire la ripresa dei consumi e degli investimenti e per consentire un deciso recupero della produzione e dell'occupazione nel prossimo periodo. del Documento di economia e finanza 2016 emerge in tutta evidenza la proposta volta a scoraggiare l'attivazione delle clausole di salvaguardia per il 2016, che avrebbero l'effetto di aumentare il prelievo a carico di cittadini ed imprese. Tale decisione rappresenta un intervento importante in grado di determinare un abbattimento significativo della pressione fiscale contemplata dal quadro tendenziale. Altro punto qualificante del Documento di economia e finanza 2016, ritenuto necessario per facilitare il processo di ripresa economica, è rappresentato dall'utilizzo della flessibilità della finanza pubblica che, insieme al complesso degli investimenti in programma, rappresenta uno snodo fondamentale per aumentare significativamente le capacità competitive del Paese. L'Italia, pertanto, si appresta ad inviare in Europa un Documento di programmazione economica e finanziaria completo, con un Programma nazionale di riforme ben delineato, dal quale ricavare le direttrici prioritarie del nostro percorso virtuoso di crescita e risanamento dei conti pubblici, con un'agenda di interventi innovativi - ben rilevabili nel PNR - di politica economica interna e una politica di bilancio responsabile, attenta all'equilibrio dei conti pubblici, che assicura la fiducia dei mercati grazie a finanze pubbliche solide, e in grado di aumentare la competitività e accrescere il potenziale di crescita nel lungo periodo. Appare però del tutto evidente, tuttavia, che senza un cambio di passo anche in Europa, l'aggancio della ripresa economica diventa per il nostro Paese più complicato. In questo percorso, si dovrà pertanto agire anche in sede europea, per impostare e concentrare l'attenzione dell'Europa proprio su tali tematiche, cioè sulla crescita, e per aprire nuovi e maggiori spazi di manovra per favorire una crescita economica sostenuta, duratura e al passo con l'andamento dei paesi maggiormente sviluppati. Ricordo che l'Annesso al Documento di economia e finanza 2016 reca la Relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, che richiede l'autorizzazione ad aggiornare il piano di rientro verso l'Obiettivo di medio periodo. Ai sensi del richiamato articolo 6, la deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza l'aggiornamento del piano di rientro è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Pertanto, l'esame del Documento si concluderà con l'approvazione di due distinti atti di indirizzo: il primo relativo alla Relazione di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, da votare a maggioranza assoluta; il secondo relativo al Documento di economia finanza, da votare a maggioranza semplice. Le proposte di risoluzione ad entrambi i documenti dovranno essere presentate entro la fine della discussione. Ricordo che i tempi della discussione sono stati ripartiti tra i Gruppi secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo.

Nell'arco di un paio di anni sono stati sequestrati e confiscati beni per miliardi di euro. Solo a un prestanome di Matteo Messina Denaro, Vito Nicastro, sono state confiscate definitivamente 43 società che operano nell'energia pulita, per un valore di 1,3 miliardi di euro; solo su Roma e dintorni, il procuratore della Repubblica Pignatone calcola un patrimonio mafioso intorno a 1,5 miliardi tra beni e denari sequestrati e in via di confisca. A Piombino, in Toscana, a fine marzo sono stati sequestrati un bar e 260.000 euro su un conto bancario intestato a un camorrista. Questi sono pochi e sparsi esempi di un conto vertiginoso. Forse oggi che parliamo di DEF e di economia, quelli che fanno finta che la legalità non sia un problema economico oggi lo capiranno. Mafie e corruzione sono un problema economico. Isaia Sales, nel suo recente libro «Storia dell'Italia mafiosa», dice testualmente che: «Una criminalità è di tipo mafioso se reinveste capitali, accumulati con l'uso della violenza, nell'economia legale, senza però mai lasciare definitivamente gli affari illegali anche quando ha messo solide radici nell'economia lecita e non si limita solo ad attività predatorie». Ecco spiegato perché nella terza sezione del DEF, a pagina 486, c'è un paragrafo dedicato al contrasto alla corruzione e alla criminalità economica, alla riforma della prescrizione dei reati e alla valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Si tratta, per la verità, i passaggi un poco sbrigativi, troppo sintetici. Denotano la consapevolezza del tema, ma non la necessaria convinzione nell'affrontarlo. Infatti non possiamo più tollerare i dati sulla prescrizione: solo nel 2013 sono stati cancellati 68.107 procedimenti davanti al GIP, 20.685 in primo grado, 21.521 in sede di appello. Non c'è solo il tema dell'impunità per chi commette reati; c'è anche lo spreco di denaro pubblico per una giustizia che gira a vuoto, non perché fannullona, ma per colpa di una legge chiamata Cirielli. Il professor Lucio Picci, professore di economia all'università di Bologna, studioso di corruzione e membro della commissione statistica della Presidenza del Consiglio, ritiene che il costo della corruzione sia largamente superiore al danno erariale dato dalle tangenti e difficile da quantificare con precisione. Tuttavia, su «Il Sole 24 Ore» si è cimentato su una stima: utilizzando come misura della corruzione un indice basato sulla percezione del fenomeno e una valutazione del suo danno economico complessivo ottenuta per mezzo di tecniche econometriche, il costo del differenziale tra costi della corruzione in Germania e in Italia è di circa 585 miliardi all'anno. Se questi fondi fossero redistribuiti agli italiani il loro reddito *pro capite* non solo aumenterebbe di 10.607 euro all'anno, ma supererebbe quello dei tedeschi di circa 1.000 euro. Sulle medesime posizioni si colloca Alberto Vannucci, ordinario di scienza della politica, recentemente intervenuto in un importante convegno nella mia città (Desio) e ascoltato a Milano qualche giorno fa dalla Commissione d'inchiesta antimafia. Vedete, colleghi, nello stesso DEF vi è una parte interessante dedicata alla cultura, alla ricerca e all'istruzione. Vi si dice, in sostanza, che per sostenere la produttività nel medio e lungo termine è necessario, tra l'altro, continuare a sviluppare il capitale umano che include il miglioramento dell'istruzione, lo sviluppo della ricerca tecnologica, la promozione della scienza e della cultura, facendone vera priorità della politica nazionale. Per fare tutte queste cose, che sono buone e giuste, occorrono risorse, investimenti, insomma spesa pubblica. Serve quindi riappropriarci delle risorse che, direttamente o indirettamente, le mafie e la corruzione ci sottraggono. Quali sono le conseguenze pratiche di questi ragionamenti? Chiedo che nella risoluzione con cui si approverà il DEF siano indicate alcuna priorità legislative e che siano collegate alla manovra di finanza pubblica: la riforma della prescrizione e la riforma del codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Solo con il formale collegamento al DEF di questi provvedimenti noi daremo la sensazione che la lotta alla corruzione e alla mafia è divenuta una priorità economica del Paese. nella Relazione al Parlamento che accompagna il DEF si evince chiaramente che la stima di crescita del PIL per il 2016 è del 1,2 ma potrebbe essere soggetta a rischi al ribasso dovuti all'incertezza relativa alla domanda interna e alla capacità delle imprese italiane di espandere le loro esportazioni in un quadro di accresciuta difficoltà economica. Noi riteniamo che i provvedimenti adottati dal Governo hanno sostenuto pochi settori, tra i quali quello delle banche e quello dell'energia fossile, privilegiando però il mantenimento delle rendite e non invece un circolo virtuoso di crescita. Il Governo non è stato capace di intraprendere azioni nell'ambito della concorrenza dei mercati e ricordo che nella mia Commissione l'esame del provvedimento sulla concorrenza è interrotto dalle note vicende legate allo scandalo Tempa Rossa

che graverà quindi sulle capacità competitive delle aziende, contribuendo a generare deflazione? Noi qui abbiamo interrotto bruscamente un circuito virtuoso di investimenti nel settore delle rinnovabili e dell'autoproduzione decentralizzata. Lo abbiamo interrotto quando era una delle poche cose che funzionava bene. Non ci sono novità in merito ad altri settori fondamentali e potenzialmente ricchi come il turismo, la cultura, il commercio e la produzione di beni di consumo tipici italiani, che non sono però sufficientemente tutelati nella loro identità di *made in Italy*. Anche nell'innovazione e nella ricerca, due capisaldi fondamentali per lo sviluppo sostenibile, siamo in forte ritardo e fanalino di coda tra i Paesi industrializzati. Invece si investono capitali in settori ormai obsoleti grazie alla svendita di un patrimonio di avanguardia senza immaginare un piano di valorizzazione e rilancio; mi riferisco al caso Versalis, che deve farci riflettere e che dobbiamo maggiormente Dobbiamo intervenire con urgenza cambiando modello di produzione, spostando gli interessi su altri settori. In particolare, ad esempio, anziché fare uscire migliaia di euro verso l'estero per soddisfare la domanda interna di energia, quindi importando energia (perché l'80 per cento con conseguenze anche per i Paesi belligeranti che ci circondano, potremmo e dovremmo investire nella riduzione dei consumi e nella produzione interna con fonti rinnovabili. Ricordiamo che l'efficienza energetica è la nostra prima vera grande fonte energetica, ma ancora non vedo la concretizzazione di quella mozione per la stabilizzazione dell'ecobonus che abbiamo votato all'unanimità due settimane fa. Se invece intraprendessimo questo cammino, libereremmo risorse pulite e favoriremmo un circuito finalmente virtuoso di progresso sociale, economico, ambientale e sanitario, con la generazione di nuova occupazione in grandi numeri, e avremmo la riduzione delle emissioni inquinanti e la tutela del territorio, che in questo momento invece sono due punti molto dolenti. Faccio notare anche quello che scrive nero su bianco l'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) che dice che «l'eventuale emergere di sorprese negative sul fronte della crescita reale e dell'inflazione metterebbe a rischio la dinamica del PIL nominale e, con essa, il percorso di abbassamento del rapporto debito/PIL». L'UPB fa notare che i numeri contenuti nel DEF, nella forchetta di possibilità, sono sempre presi nella stima più rosea: non c'è spazio di manovra in caso di un qualsiasi compromesso. Di fatto, il Governo ha imperniato il DEF su una previsione di crescita del PIL che corrisponde all'estremo più alto della forchetta, quindi, le conseguenze negative, che non si possono escludere, lo inficerebbero assai.

smonta il DEF e taglia le stime di crescita previste per il 2016 e 2017, affermando testualmente che: «La crescita è stata più lenta del previsto in Italia».

Signora Presidente, nel mio breve intervento mi occuperò, in modo particolare, del problema della sanità. fuori dubbio che il Sistema sanitario nazionale, rispetto ad altri sistemi internazionali, si evidenzia in modo particolare per il problema dell'universalità: abbiamo sempre considerato la salute un bene primario e, quindi, spetta allo Stato, sulla base delle tasse che i cittadini pagano, fornire dei servizi notevolmente adeguati. Un interessantissimo documento dell'Istituto superiore di sanità ci dà alcuni dati che sono, secondo me, la premessa indispensabile per capire e giudicare l'atteggiamento del Governo relativamente al problema della sanità, soprattutto per quanto riguarda la disponibilità di risorse, i costi e l'assetto strutturale di questo nostro Paese.

Purtroppo si è evidenziato che, rispetto all'aumento delle patologie, all'invecchiamento della popolazione e alla riduzione delle risorse, la sostenibilità del sistema, a breve, potrebbe avere delle problematiche.

per la ristrutturazione delle strutture ospedaliere perché, così come sono combinate, soprattutto in alcune realtà del Paese, diventano assolutamente ingestibili e improduttive. Per non parlare, poi, del problema del personale:

(senza citare i blocchi contrattuali che si sono avuti). Questo cosa comporta in modo particolare? Che il divario esistente nelle varie Regioni d'Italia si fa sempre più profondo.

1.530 nel 2018 e 1.589 nel 2019), la dice lunga su quelli che sono i comportamenti di questo Governo relativamente alle premesse e alle conclusioni. se le premesse sono condivisibili - e le premesse sono nel parere espresso dalla 12a Commissione - mi pare che le proposte che vengono fatte relativamente al problema della sanità vadano in senso opposto;

di conseguenza, si registrano, proprio sul piano degli strumenti programmatori riguardanti le opere pubbliche e le infrastrutture, le più immediate novità. Da questa edizione del DEF viene meno, infatti, l'allegato infrastrutture, che, a partire dell'anno successivo, sarà sostituito da due nuovi strumenti programmatori. Il primo, il Piano generale dei trasporti e della logistica in realtà costituisce per noi una vecchia conoscenza. Inaugurato dall'allora ministro Bersani come strumento ordinario di pianificazione delle opere pubbliche, durò però una sola stagione. Con il cambio di Governo e con l'esperienza del secondo Governo Berlusconi, si aprì infatti la stagione della legge obiettivo: un periodo che oggi valutiamo, al netto di tutte le facili polemiche sulle realizzazioni e sugli obiettivi disattesi, infruttuoso proprio dal punto di vista della pianificazione e della strategia di sviluppo del Paese. Non è un caso che il limite più grave introdotto con la legge obiettivo sia stato proprio il sistema corruttivo, che ad ogni livello essa ha tollerato e favorito. Oggi, a partire da questo DEF e con quelli che seguiranno, torniamo così alla centralità degli strumenti ordinari di pianificazione delle opere pubbliche. Infatti, è solo da una seria programmazione, che sia davvero in funzione delle nuove esigenze di mobilità delle persone e della maggiore efficienza logistica per le merci, che può derivare una corretta e trasparente selezione delle priorità in ragione dell'effettiva disponibilità delle purtroppo scarse risorse pubbliche. Il secondo strumento programmatorio è il Documento di programmazione pluriennale. Si tratterà di uno strumento triennale più operativo, con relativo aggiornamento annuale delle opere programmate per le quali viene prevista l'effettiva realizzazione; uno strumento, quindi, specifico di selezione delle priorità per l'azione di Governo. Anche le direttrici contenute nell'allegato di questo DEF, che potremmo definire di transizione, sono chiare e per noi assolutamente condivisibili. In primo luogo, la politica dei valichi e dei trafori di connessione ai corridoi transeuropei: una partita sfidante per il nostro Paese in termini di competitività di sistema con gli altri Paesi membri dell'Unione europea, e riguardante l'efficientamento della nostra rete logistica sia per le infrastrutture materiali, che per quelle immateriali. Da un lato, ferrovie e autostrade che superino le barriere fisiche alpine, che hanno da sempre determinato la condizione di insularità del nostro Paese; dall'altro, le procedure digitali che consentano di abbattere, già oggi con più facilità rispetto al passato, la burocrazia, e con essa i tempi morti di stanziamento delle merci, come avviene, per esempio, nei porti. In secondo luogo, vi è finalmente anche la consapevolezza, da parte di questo Governo, che, se la partita si gioca sui valichi alpini, questa sfida può essere vinta soltanto se vengono organizzati meglio, dal punto di vista infrastrutturale, anche i nostri mercati di produzione e di consumo. Dalla connessione dei distretti produttivi agli scali portuali e aeroportuali vi è una richiesta infrastrutturale diffusa di collegamento con le principali arterie ferroviarie dell'Alta Velocità e con quelle autostradali. Infine, l'elemento che più di altri contraddistingue l'innovazione che la nuova stagione intende perseguire è l'attenzione per i centri urbani e le grandi aree metropolitane. Qui il Governo intende intervenire con un ricco programma di opere ferroviarie, dalle metropolitane alle tramvie, che vogliono rappresentare in concreto la cura del ferro annunciata. E, a corredo di questi, ci sono anche progetti di una mobilità più intelligente e flessibile, che costituiscono la cifra di una nuova sensibilità attenta tanto all'efficienza dei trasporti quanto alla qualità della vita. Si tratta di un programma che non ha eguali per dotazione di piste ciclabili e progetti di connessione tra le varie modalità di trasporto, per realizzare una compiuta integrazione modale; insomma, la promozione su vasta scala di una modalità di trasporto più consona e adeguata in funzione della distanza di percorrenza. Lo stato di efficienza di un Paese, di un grande Paese come il nostro, non si risolleva dalla crisi materiale di questi anni e da quella morale degli anni precedenti in un attimo. Occorrono metodo e rigore al servizio di una strategia chiara ed efficace, in funzione dell'interesse generale. In questo senso, i presupposti contenuti nell'Allegato al DEF ci fanno ritenere che una stagione di cambiamenti positivi si sia finalmente aperta e che questa prospettiva debba essere perseguita con convinzione e tenacia. Noi siamo certi, in questo senso, che i risultati già in corso verranno quindi a maturazione. il DEF, il Documento di economia e finanza, dovrebbe rappresentare un atto importante per l'azione di Governo. Dovrebbe infatti contenere impegni volti al consolidamento delle finanze pubbliche e dovrebbe definire gli interventi volti al raggiungimento di obiettivi come la crescita, la produttività e l'occupazione. Quindi, in apparenza, questa discussione dovrebbe rappresentare un momento importante. Nella realtà, purtroppo, questo Documento

lo saranno probabilmente anche quest'anno, soprattutto su alcuni valori fondamentali, come la previsione del PIL. Ricordiamo che l'anno scorso per la prima volta - è stata forse l'unica eccezione alla regola - è stata fatta una previsione della crescita del PIL sostanzialmente

Quest'anno il Governo prevede una crescita del PIL dell'1,2 per cento, a fronte di previsioni del Fondo monetario internazionale e dell'OCSE che invece segnano un più uno per cento nella migliore delle ipotesi. Da questo punto di vista, il Governo ha messo in evidenza un'inversione di tendenza che ritiene strutturale ed importante. È vero che negli anni passati il PIL non è mai cresciuto, anzi aveva un segno negativo, e che nel 2015 per la prima volta c'è stata questa inversione di rotta. È giusto però anche ravvisare e ricordare che l'Ufficio parlamentare di bilancio definisce la crescita del PIL italiano «anormalmente» lenta. Questa è l'espressione che è stata utilizzata, perché, se c'è un +0,8 per cento dell'Italia, allo stesso tempo ravvisiamo un

il nostro e la sua situazione economica non facile, riscontra una crescita del PIL che è nettamente superiore a quella italiana e ci fa rimanere una delle ultime ruote del carro della crescita e della ripresa economica,

che risulta sempre più inutile per una programmazione certa e per ottenere, anche da parte del Parlamento, un voto consapevole sulle proposte di risoluzione che verranno presentate. Ravvisiamo altri punti deboli, uno dei quali legato alle privatizzazioni. Nel 2015 sono state fatte privatizzazioni per un valore di 6,5 miliardi di euro, pari allo 0,4 per cento del PIL. Teoricamente, queste privatizzazioni dovevano portare a una riduzione del debito pubblico, perché questo dovrebbe essere lo scopo, l'intento, il fine

altresì la spesa senza controllo per l'ospitalità dei clandestini nel nostro Paese, che sarà in aumento anche quest'anno,

a grave danno soprattutto della nostra sanità, che è uno dei nostri patrimoni più importanti. Il Governo, quindi, impone agli altri ciò che non è in grado di fare e di imporre a se stesso. La riduzione dei costi dell'apparato statale non è stata attuata né avviata e si gettano le responsabilità solo sulle spalle dei poveri amministratori locali che sono in grave difficoltà nel tenere insieme le necessità di non aumentare la pressione fiscale e di garantire...

Signora Presidente, onorevoli colleghi, ormai dovrebbe essere chiaro che ai parlamentari nazionali dell'area euro è demandato sempre di più il ruolo di meri certificatori di vincoli e imposizioni decisi altrove. Vincoli ed imposizioni che non rispecchiano affatto le effettive e peculiari esigenze socio-economiche di ciascun Stato, anche perché il disegno di dotare l'Europa di un effettivo mercato unico e di creare la cosiddetta Europa dei popoli è rimasto praticamente sulla carta e nelle intenzioni dei Trattati. Il Documento di economia e finanza, che sia quello del 2015 o del 2016, ne è la prova più evidente, perché, per quanti miglioramenti possano essere apportati a questo testo, l'unico gesto sensato sarebbe quello di respingerlo *in toto* è pieno di rimandi e rinvii, cifre basate su ottimistiche previsioni future; cifre indefinite in attesa di tempi migliori e di una ipotetica crescita e previsioni totalmente inattendibili, pur di cercare benevolenza e consensi a Bruxelles o forse, semplicemente, per seguire la falsariga dei *Diktat* europei, piuttosto che proporre programmi di politica economica efficaci e coerenti con l'attuale situazione economica italiana per il rilancio della domanda interna, investimenti e occupazione. Appare ormai chiara la distanza dell'Italia rispetto alla crescita media europea, con un tasso di occupazione che rimane stabilmente al di sotto della suddetta media. un Documento incentrato, fin dall'inizio, non solo su politiche di riduzione di un debito che effettivamente i cittadini non hanno contratto, ma attraverso il quale, addirittura, si pensa di ridurre il rapporto debito-PIL mediante la cessione di proprietà pubblica: la solita menzogna che si racconta per motivare ogni grossa privatizzazione attuata finora. Occorre ricordare come la protezione assoluta dei diritti sociali oggetto delle conquiste della nostra civiltà sia oggi subordinata al perseguimento dell'obiettivo della stabilità dei prezzi. Sacrifici e ancora sacrifici vengono imposti agli italiani in nome del pareggio di bilancio, metastasi antistorica, dissennatamente inoculata nella nostra legge fondamentale. Il DEF non dà risposte alle reali e molteplici emergenze sociali del Paese. Onorevoli colleghi, il costo che ci impone l'Europa è ineludibile: svalutare i diritti di lavoratori, pensionati, malati e studenti, con effetti più che proporzionali sull'economia reale, che si vorrebbe rilanciata, mentre imprese che un tempo erano il nostro fiore all'occhiello vengono comprate da chi si vuole appropriare della nostra storia o da chi vuole sbarazzarsi, ora, di pericolosi concorrenti. Come il tentativo di smantellare il sistema sanitario pubblico per il profitto dei privati, rimanendo in linea con le politiche di un Governo che ha portato al risultato che molti cittadini hanno rinunciato a curarsi per l'aumento del *ticket* e le interminabili liste d'attesa. Per il 2016 erano previsti 117,6 miliardi di euro dal DEF precedente del 2013, calati poi, invece, a 113,4 con il DEF 2015, per arrivare a un finanziamento reale di 111 111 miliardi, comprensivi di 800 milioni di euro per i nuovi LEA. Stiamo demolendo sistematicamente la più grande conquista sociale dei cittadini italiani: un servizio sanitario pubblico, equo e universalistico, da difendere e garantire alle future generazioni. Andando nello specifico e confrontando gli attuali dati con quelli contenuti nel DEF del 2015, l'attuale coalizione di Governo sarà soddisfatta per aver

una preoccupante sovrastima delle imposte dirette per ben 6,5 miliardi di euro, compensata parzialmente da un incremento delle imposte indirette dovute essenzialmente all'ampliamento della pratica del *reverse charge*. Dal lato delle uscite vi è stata una diminuzione delle retribuzioni dei dipendenti della pubblica amministrazione per 3,1 miliardi di euro, variazione piuttosto inspiegabile visto che il numero di unità di lavoro non è diminuito. Anche tenendo conto del fatto che il miliardo di euro previsto per la «buona scuola» non sia stato tutto di competenza del 2015, questo calo, a parità di forza lavoro, rimane inspiegabile. In realtà, il dubbio è che il sostanziale azzeramento dei pagamenti delle ore straordinarie per gli uffici non di *staff* e il forte taglio alle componenti del salario di produttività abbiano contribuito a questo ridimensionamento assolutamente controproducente in un'evidente crisi di domanda aggregata. Tutto ciò fa sì che grandi e potenti *lobby* riescano a rendere più debole l'apparato pubblico in modo da impadronirsi dei suoi mezzi e competenze, sovente a prezzi di comodo. D'altronde, come fidarsi di un Governo che si fa portavoce delle *lobby* delle trivellazioni in mare e il cui Presidente del Consiglio lancia moniti a favore dell'astensionismo per un *referendum* al riguardo? di una politica ambientale europea che sostiene la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio come pratica sicura e che invece è una tecnologia immatura, costosa e rischiosa, che più che porre un argine alla emissione di gas serra è una giustificazione per costruire nuove centrali a carbone? Come quando si parla di energia rinnovabile e poi si assiste alla proliferazione incontrollata delle centrali a biomasse che, seppur in linea di principio non producono CO2, tuttavia portano ad un incremento delle emissioni di inquinanti in atmosfera, determinando concretamente un peggioramento della qualità dell'aria. Posso pertanto concludere che solo la fortuna ha portato l'entità delle entrate e delle uscite a compensarsi, non certo per una reale capacità del Governo nel pianificare e programmare i fenomeni economici a supporto delle reali Abbiamo sacrificato ogni cosa sull'altare di una integrazione europea che ha costi insostenibili sotto il profilo economico, sanitario e umano. Ebbene, il peggiore augurio che il Fondo monetario internazionale ha formalizzato è sciaguratamente e finalmente arrivato. Grazie a questa ulteriore manovra, la compressione dei diritti del cittadino ritrova un'interpretazione tra le più cupe del nostro millennio: dobbiamo chiedere ai nostri cittadini cittadini ogni sacrificio, privandoli di ogni speranza, allungando irragionevolmente i tempi del pensionamento, ma soprattutto scoraggiando in ogni modo quelle legittime aspettative di vita che sarebbe stato necessario coltivare e incoraggiare.

Signora Presidente, colleghi, nel mio breve intervento mi concentrerò solo su alcuni aspetti del DEF affrontati nell'8a Commissione, di cui faccio parte, faccio parte, relativamente alle infrastrutture di trasporto e della logistica che, a mio avviso, rappresentano uno dei nodi più importanti dell'azione di governo, che determinerà in modo consistente il successo o no dell'intera strategia economico-finanziaria che ha come obiettivo primario la crescita economica e occupazionale del nostro Paese. Dopo questi due anni di Governo Renzi, il 2015 si è chiuso con il segno positivo, che non vedevamo da anni. Abbiamo fatto molta fatica per invertire la tendenza ed ottenere lo 0,8 per cento Siamo riusciti a rimuovere solo alcuni degli ostacoli che hanno bloccato, in questi anni, il sistema produttivo del Paese e il suo sistema politico istituzionale. Per sbloccare il sistema Paese abbiamo messo in discussione, ora in particolar modo, quei mostri sacri che hanno regolato le politiche economiche negli ultimi dieci anni: uno di questi è il Patto di stabilità, che ha prodotto il crollo degli investimenti pubblici, fino quasi al loro dimezzamento. Lo sblocca Italia 2014, il primo allentamento del Patto di stabilità dei Comuni e l'accelerazione di spesa dei fondi della Unione europea hanno permesso all'Italia, nel 2015, di invertire la tendenza e tornare alla crescita, anche nel settore degli investimenti (anche se flebile). Le misure contenute nella legge di stabilità 2016 - mi riferisco alla clausola investimenti, alle maggiori risorse ANAS e Ferrovie, all'addio al Patto nei Comuni - hanno il compito di far ripartire su tutto il territorio nazionale i cantieri di quelle opere pubbliche attese e rinviate per anni: ferrovie, scuole, strade, musei, biblioteche, superando così il *gap* infrastrutturale che ci separa dagli altri Paesi europei e nello stesso tempo dando impulso alla ripresa economica a partire dal settore edile, che ha visto perdere negli anni centinaia di migliaia di posti di lavoro. I dati positivi di produzione industriale registrati nei primi mesi del 2016 lasciano prefigurare una nuova accelerazione del prodotto interno lordo nei prossimi trimestri. In linea con tali andamenti, il DEF prevede per il 2016 un incremento del PIL pari all'1,2 Nello scenario programmatico, l'accelerazione della crescita proseguirebbe anche nel biennio successivo, grazie ad una politica di bilancio orientata al sostegno dell'attività economica e dell'occupazione, con interventi finalizzati ad un miglioramento della competitività

peraltro frammentata e disorganica, e di un'assenza di pianificazione e programmazione. Per lo sviluppo del sistema nazionale dei trasporti sarà fondamentale perciò dare attuazione sia alle misure previste nel Piano nazionale degli aeroporti, predisposto pochi mesi fa, sia agli investimenti per la rete ferroviaria che costituisce una priorità - e voglio io sottolineare: una priorità - del Governo in materia di trasporti. Nell'ultimo biennio sono stati stanziati 17 miliardi di euro di risorse aggiuntive, 9 dei quali già destinati all'aggiornamento, per il 2015, del contratto di programma con Rete ferroviaria italiana (RFI). Soldi finalizzati a migliorare la sicurezza e le tecnologie per la circolazione dei treni, potenziare il trasporto passeggeri nelle aree metropolitane, regionali e lungo i corridoi europei e per il miglioramento del trasporto merci. Gli altri 8 miliardi saranno oggetto dell'aggiornamento del contratto per il 2016. Con riferimento alla rete stradale, il piano pluriennale di ANAS 2015-2019, rivolto prevalentemente al rafforzamento degli *asset* infrastrutturali strategici del Paese, al miglioramento degli accessi in città e al potenziamento dei collegamenti intermodali, prevede investimenti su più di 3.600 chilometri di strade per un importo complessivo di 15 miliardi di euro, di cui per il completamento di itinerari, 7,3 miliardi destinati alla manutenzione straordinaria e 1,4 miliardi per le nuove opere, principalmente in corrispondenza dei nodi urbani. Il rafforzamento infrastrutturale dei nodi urbani principali del Paese rappresenta una scelta strategica del DEF. Infatti, se prendiamo a riferimento le principali 8 città metropolitane vediamo che lì si trovano i poli industriali e manifatturieri più importanti importanti e significativi, dove è concentrato il 31,9 per cento del valore aggiunto del settore industriale e il 30 per cento di quello manifatturiero. Dotare questi nodi di infrastrutture materiali e immateriali adeguate significa perciò non solo garantire una migliore accessibilità a milioni di persone, ma anche e non di meno, portare un contributo al rafforzamento dei nostri distretti manifatturieri e perciò alla diminuzione della disoccupazione. Presidente, onorevoli colleghi, nessuno può negare in quest'Aula che il quadro economico internazionale, nonostante le previsioni più ottimistiche registrate a inizio 2015, sia peggiorato nel corso della seconda parte dello scorso Tutto ciò ha rappresentato un motivo di freno per la crescita della nostra economia, che comunque è riuscita a conseguire una crescita che si attesta allo 0,8 per cento: a taluni potrà sembrare un dato deludente, ma costituisce pur sempre una crescita. Non dobbiamo dimenticare infatti che le previsioni economiche non si palesano mai esatte, soggette come sono a variabili non facilmente ponderabili, come per esempio l'entrata in recessione dell'economia di alcuni Paesi emergenti oppure le conseguenze psicologiche ed economiche degli attacchi terroristici accaduti recentemente o, ancora, le turbolenze finanziarie che hanno interessato l'economia degli Stati Uniti d'America o la forte discesa del prezzo del petrolio. Per non parlare dell'emergenza migranti, che ha rivelato tanti punti di debolezza della strategia europea nell'affrontare tale questione. Tutti fattori che giocoforza hanno determinato la revisione degli obiettivi del Governo anche sul Documento di economia e finanza del 2016. Per cui nessuno scandalo, cari colleghi, se il tasso di crescita previsto nel DEF per il 2016 scende all'1,2 per cento rispetto al dato dell'1,6 per cento previsto nella Nota di aggiornamento precedente. Si tratta di una giusta previsione prudenziale che, come sottolineato giorni fa dal Presidente del Consiglio, depone per un atteggiamento di responsabilità e di serietà da parte del Governo. E ciò anche perché comunque si continua a pensare che la domanda interna reggerà e che le imprese italiane saranno capaci di espandere le loro esportazioni. Quindi, al di là delle critiche, è incontrovertibile che l'economia italiana cresce, e che tale crescita si accompagna al miglioramento continuo delle finanze pubbliche, sia in termini di *deficit* che di debito. Il tasso di occupazione è cresciuto e anche l'andamento

Anche il debito scenderà e anche in questo caso, prudenzialmente, è stata prevista una discesa meno verticale, ma l'inversione di tendenza ci sarà: il rapporto debito/PIL scenderà al 132,4 per cento quest'anno e al 130,9 per il dato che dobbiamo comunque prendere in considerazione è che a fronte di questo scenario il Governo ha annunciato che non ci saranno manovre correttive, anzi è previsto che la pressione fiscale nel 2016 scenderà al 42,8 per cento, con una diminuzione di 0,7 punti e questo accadrà anche considerando gli effetti che il *bonus* di 80 euro avrà sul reddito netto dei lavoratori. D'altronde, per continuare la politica di sostegno alla crescita coniugandola con il rafforzamento e risanamento della finanza pubblica, qualche scelta importante va pure fatta, al pari con l'assunzione di qualche forte responsabilità e mi pare che in questo senso si stia procedendo. Certamente l'obiettivo del rapporto *deficit*/PIL del rapporto *deficit*/PIL all'1,8 per cento nel 2017, rispetto all'1,1 per cento delle previsioni dello scorso autunno, lascia supporre una richiesta di flessibilità di 0,7 punti di PIL, pari a 11 miliardi, e proprio su questo punto si sono scatenate fior di polemiche, dal momento che molti dubbi sono stati sollevati sulla possibilità di ottenere ulteriore flessibilità dall'Europa. Invece, cari colleghi, va detto chiaramente che il cammino delle riforme avviato dal Governo e sostenuto dal Gruppo AL-A consente di richiedere e utilizzare ulteriore flessibilità, per cui la previsione di un 1,8 per cento di *deficit* nel 2017 è del tutto compatibile con lo scenario europeo e cioè con lo specifico riferimento a quelle circostanze eccezionali che riguardano il deterioramento marcato del contesto internazionale. Su questo punto si sono scatenate, come abbiamo potuto sentire anche in quest'Aula, esternazioni di scetticismo e di preoccupazione. Tuttavia, cari colleghi, mi permetto di farvi riflettere sul fatto che il percorso riformatore del Governo consente al nostro Paese di poter ventilare una simile richiesta di flessibilità, in quanto la situazione italiana per quanto riguarda i conti pubblici è migliore rispetto a quella di altri Paesi, sia per effetto delle riforme, che per gli investimenti. Se fossimo la Francia, forse queste perplessità sarebbero fondate, ma nel nostro caso sarei cauto nel dare credito ai pessimisti. La verità innegabile è che l'Italia è stata immersa per anni in una crisi senza precedenti che ha evidenziato i forti problemi strutturali del Paese; pertanto, a causa di questa situazione, è normale che lo sforzo d'inversione di una tendenza visibilmente grave e che ha impattato su tutte le fasce della popolazione debba essere necessariamente prolungato nel tempo. Non è possibile, cioè, evocare ricette miracolistiche che hanno il sapore di essere state create da apprendisti stregoni. All'interno del Documento che stiamo esaminando sono presenti, invece, gli ingredienti fondamentali per una strategia realistica di ripresa del nostro Paese: continuare nella riforma strutturale dell'Italia stimolando gli investimenti, sia privati che pubblici; continuare a stimolare la creazione di nuova occupazione, oltre a quella che è stata incrementata nel corso del 2015; consolidare gradualmente le finanze pubbliche, in maniera tale che venga ridotto il rapporto tra debito e PIL; la riduzione progressiva della pressione fiscale; l'individuazione e la lotta agli sprechi accompagnata da una maggiore efficienza della giustizia civile e dalla razionalizzazione della spesa e dell'attività della pubblica amministrazione; continuare nelle azioni per aumentare la competitività del sistema Italia. Tutte queste azioni guardano certamente al medio e lungo periodo, ma è questo l'orizzonte temporale a cui dover fare riferimento per superare quei *gap* storici che hanno determinato fragilità determinato fragilità del nostro sistema economico che la grande crisi, esplosa nel 2008, ha messo in evidenza con drammatica crudezza. Tuttavia, noi vogliamo mostrarci fiduciosi, convinti come siamo che la vera ripresa è fatta di sforzi, di coraggio, di fatica, di piccoli e costanti passi che ci traguardino verso l'obiettivo più grande che è quello di migliorare la qualità della vita degli italiani. *(Applausi l'unica cosa che si comprende benissimo in questo DEF - tanto per cambiare - è che c'è un ulteriore attacco al mondo del lavoro,

In questo DEF non c'è ombra del reddito minimo garantito, eppure le nostre famiglie si stanno impoverendo: ormai 10 milioni di famiglie vivono nella povertà.

Le affermazioni fatte da colui che voi definite «il professor» Ichino sono agli atti: vi invito a riflettere. E mi rivolgo soprattutto a quella parte della politica che pensa che il mondo del lavoro non possa essere ridotto a merce.

Una ripresa che è assente, tanto è vero che la crescita delle disuguaglianze e della povertà non si ferma e il Mezzogiorno d'Italia è sempre più il Sud dell'Europa. Un altro grande assente nel DEF è la politica economica. Il Governo si è affidato alla favorevole congiuntura internazionale e alle riforme strutturali di stampo neoliberista che, sino ad ora, hanno lasciato un certo dissapore. Tassi d'interesse e petrolio così basso non dureranno ancora per molto. Sempre il Governo continua a cavalcare l'onda europeista aderendo all'approccio di bilancio europeo, caratterizzato da tagli lineari sulla spesa pubblica, sostenendo i profitti e riducendo salari e protezioni sociali. Tutto ciò al fine di raggiungere il fantomatico pareggio di bilancio che, nonostante gli sforzi che i cittadini sono stati chiamati ogni giorno a sostenere, è stato ancora una volta posticipato, con la previsione di essere raggiunto nel 2019. Nel DEF la spesa sanitaria nel 2019 scenderà al 6,5 per cento del PIL, cioè al di sotto del livello di rischio per la salute indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. A ciò si aggiungano gli interventi su previdenza e Stato sociale. Allo stato attuale, il DEF esclude interventi a sostegno della flessibilità in uscita, in materia di pensioni, ed esigue sono le risorse economiche stanziate per nuclei familiari con figli minori. Si continua a percorrere la strada che porta alla riduzione del *deficit* e del debito pubblico in maniera più attenuata, rimanendo aderente alla linea della cosiddetta austerità flessibile. È evidente l'incapacità di destinare le poche risorse disponibili verso il vero sviluppo economico che per noi non è la crescita, ma il benessere ed il progresso culturale e sociale di un popolo. Nel DEF 2016 non c'è alcuna traccia di valutazione dell'indicatore Benessere Equo e Sostenibile (BES). Si è talmente conservatori che si fatica a svincolarsi dai soliti parametri economici? Ci auguravamo che PIL e BES potessero camminare insieme, in modo da permettere un confronto nuovo sulla crescita del Paese, anche dal punto di vista della qualità della vita e non solo in base agli indicatori economici sempre più obsoleti. Stiamo parlando in fondo di indicatori come salute, istruzione e formazione, lavoro e conciliazione dei tempi di vita, benessere economico, relazioni sociali, sicurezza, ambiente, ricerca e innovazione, qualità dei servizi. Insomma, non stiamo parlando solo ed esclusivamente di portafogli industriali, di valori di mercato, di azioni in borsa. Come può questo Governo fondare la sua strategia politica quando, al lievissimo miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie, non corrisponde però una riduzione dell'indicatore di grave deprivazione materiale? Tale indicatore rileva la quota di persone in famiglie che sperimentano sintomi di disagio, come quello di non potere riscaldare adeguatamente la propria abitazione o non sapere come sostenere una spesa imprevista come potrebbe essere una malattia improvvisa. Noi rimaniamo fermi nell'idea che il Governo debba cambiare direzione, puntare a porre in essere investimenti pubblici seri e mirati per generare occupazione stabile e ad impegnare le proprie risorse per diminuire le diseguaglianze sociali presenti in tutto il territorio. Tutto ciò non potrà che tenere conto anche di interventi volti a riqualificare la spesa pubblica, garantendo il livello dei servizi essenziali al cittadino. inoltre, evitare la svendita delle quote del patrimonio nazionale, nonostante il Governo si ostini a perseguire la strada delle privatizzazioni per ridurre il debito. Quando sarete capaci di inserire nei documenti di bilancio e di programmazione economica non la solita clausola di salvaguardia, ma la salvaguardia della nostra felicità, allora sì che questa Italia potrà ricominciare a parlare di ripresa, di rilancio, di risveglio e, quindi, di una nuova stagione di vita democratica e sociale.

appare un dato estremamente preoccupante, contrariamente a quanto detto dal relatore nel suo intervento iniziale. Si legge proprio che l'Italia non cresce perché decresce tutto il resto del mondo.

Di conseguenza, l'Italia non può che essere un Paese al traino: se gli altri vanno bene, andiamo benino anche noi; se gli altri vanno male, noi, anziché cogliere questa opportunità per fare un passo in avanti e diventare trainanti, ci fermiamo.

Con quello che c'è scritto nel DEF però, questo non potrà mai accadere, a meno che gli altri Paesi trainanti, come gli Stati Uniti o i Paesi asiatici, non si riprendano e, di conseguenza, si portino dietro l'Italia. Il Documento economico e finanziario non può quindi non tenere conto del fatto che l'Italia è un Paese secondo e non un Paese primo.

si evidenzia come non ci sia un progetto di valorizzazione. È vero che, per la prima volta, quantomeno si prova a tracciare una strategia di sviluppo attraverso due strumenti: quello che nel DEF viene individuato come Piano generale dei trasporti e della logistica (che dovrebbe contenere le linee strategiche per la modalità delle persone e delle merci) e il Documento pluriennale di pianificazione, che attesta gli interventi relativi al settore dei trasporti e valuta meritevoli questi o quegli altri. In linea di massima, iniziare a pensare in un DEF a una programmazione che porti a uno sviluppo del Paese compiuto è certamente cosa corretta, ma bisogna vedere come si declinano i piani di sviluppo. Nella pagina successiva, infatti, si evidenzia come si arriva a una valutazione per scegliere gli gli investimenti da fare e in quali contesti, cioè attraverso gli strumenti di valutazione quantitativa, che vengono successivamente individuati nel SIMPT (il Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti). Ci

di passeggeri e merci e delle offerte - che siano attraverso ferro, gomma, trasporto navale oppure aereo - si possa arrivare a decidere dove indirizzare i finanziamenti e realizzare le opere. attraverso questo sistema, in assenza dei giusti correttivi, che cosa si può verificare? C'è domanda e offerta dove c'è sviluppo e, quindi, dove c'è più domanda ci sarà più offerta; dove non c'è domanda, e cioè in aree orograficamente compromesse (Calabria, Molise, Abruzzo, Sicilia, Sardegna, Liguria), essendoci meno domanda, ci sarà meno offerta. La responsabilità, all'interno del DEF, del Governo e dello Stato negli investimenti in questi settori è estremamente delicata, perché proprio con l'atto del Governo

Laddove andremo a privatizzare, è chiaro che la finanza e i privati non potranno investire se non in settori dove ci sia una corretta e importante remunerazione del capitale. Quindi, tratte importanti già sviluppate verranno attenzionate particolarmente dagli investitori e dai capitali. Se non ci sono dall'altra parte un correttivo e una lungimiranza, da parte del Governo e dello Stato, di investire in aree meno organizzate, meno infrastrutturate e con minori potenzialità, si verificherà un aumento del *gap* infrastrutturale tra Nord e Sud, ma soprattutto - voglio dire di più - tra aree sviluppate e aree sottosviluppate - e non intendo semplicemente Nord e Sud ma anche, come dicevo prima, aree orograficamente compromesse - che determinerà una situazione di economia a una velocità da una parte del Paese e di un'economia rallentata dall'altra parte. Nell'avviarmi alla conclusione vorrei solo sottolineare che, mentre in precedenza al DEF veniva allegato il piano delle infrastrutture, che magari si modificava di anno in anno e forse poi diventava pure il libro dei sogni,

Torino interconnessione, metropolitana di Torino, Milano-Monza metropolitana, linea 4 di Milano, tranvia di Firenze, servizio ferroviario‑metropolitana di Bologna. Il resto sono qualche chicca al Sud, alcune in Sicilia, un'opera in Sardegna e qualcuna da altre parti. È evidente che, se manteniamo come *asset* strategico queste 25 opere, privatizziamo e assegniamo ai privati la realizzazione di opere nuove

il DEF è un documento sempre ricco di dati e di stimoli, un documento complesso, come sempre. È quindi con spirito costruttivo, e annunciando il mio voto favorevole che, nei cinque minuti

abbiamo messo risorse straordinarie e irripetibili sul tema del lavoro. I risultati del 2015 sono positivi, ma certamente non altrettanto straordinari come l'impegno economico: 0,8 per cento in meno di disoccupazione. negativi del primo trimestre 2016 dimostrano che il ruolo trainante della decontribuzione era centrale e che non è stata assolutamente fondamentale l'abolizione dell'articolo 18 per i contratti a tempo indeterminato a tutela crescente nella seppur lieve crescita dell'occupazione. Sullo stesso tema, non è pervenuta ancora l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Abbiamo poi la questione dei *voucher*, che rischia, se non si apportano correttivi, di diventare una vera e propria vergogna nazionale. C'è il tema della povertà, con oltre 4 milioni di italiani che sono sotto la soglia di povertà assoluta. C'è la riforma del lavoro, con la quale si era arrivati correttamente ad abolire lo strumento della cassa integrazione in deroga, che era stato sicuramente usato usato non al meglio nel passato. Oggi, però, in assenza di una complessiva revisione degli strumenti degli ammortizzatori sociali, ci troviamo in una situazione per cui, nel solo Piemonte, circa 100.000 ex lavoratori nel 2016 non avranno più alcuna copertura. il tema della flessibilità in uscita sulle pensioni. Tutto questo richiama la fragilità della ripresa, e non solo per una crescita del PIL da "zero virgola". Appare necessario in una dimensione europea - sempre più necessario - un piano straordinario per gli investimenti; senza investimenti sani non si crea occupazione. Il Governo ha scelto gli stimoli alla domanda interna come risposta alle difficoltà sul commercio internazionale anche delle nostre esportazioni. I dati confermano una positività dell'intervento degli 80 euro, mentre difficilmente ciò avverrà, nel quadro del sostegno ai consumi interni, per l'abolizione della TASI e dell'IMU sulla prima casa in modo indiscriminato. Assistiamo, infatti, a un impoverimento dei dipendenti pubblici, al sesto anno senza contratti. Meglio sarebbe stato investire una quota di quella riduzione, un miliardo o un miliardo e mezzo, su rinnovi del pubblico impiego e anche su nuove assunzioni qualificate. Il debito pubblico, nell'obiettivo del 2016, cala dello 0,3. È a rischio - lo sappiamo tutti - se solo il PIL avesse una piccola deviazione negativa sulle previsioni. Continua, quindi, a essere un macigno sul sentiero della ripresa e della crescita. Qui c'è un tema che vorrei sottolineare, la lotta all'evasione. Nel 2015 sono stati raggiunti buoni risultati, ma fatico a condividere alcuni alcuni toni trionfalistici che ho letto. Occorre lavorare con più forza sul piano della prevenzione - si notano, ad esempio, i risultati positivi dello *split payment* - e non sul fronte della repressione. Da questo punto di vista, c'è ancora povertà di idee. La collega Guerra, nel corso dell'esame della legge di stabilità 2016, insieme a molti di noi, sul fronte della lotta all'evasione IVA - e ricordo che vale 40 miliardi - ha proposto la trasmissione in forma telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di interesse fiscale

siamo d'accordo sulla sterilizzazione, ma vi sono dubbi sulla genericità della copertura. Fin da oggi deve essere chiaro che riteniamo inaccettabile un'ulteriore manovra punitiva nei confronti degli enti locali (in particolare delle Regioni),

per aumentare la produttività che veda protagonisti i tre attori - Governo, imprese e lavoratori - e con una lotta senza quartiere a evasione, elusione e corruzione endemica. Possiamo farcela, ma dobbiamo avere maggiore umiltà di ascoltare, valutare e confrontarci e, se del caso, correggere, mai dimenticandoci che che il riformismo è anzitutto pragmatismo e non un'ideologia.

Nel campo dell'alta formazione le immatricolazioni sono diminuite un po' in tutta Italia - questo è vero - ma negli atenei meridionali la diminuzione è stata pari a quasi il doppio rispetto a quelle delle altre Regioni d'Italia. al diritto allo studio e alle borse di studio, nelle Regioni meridionali il 35 per cento degli aventi diritto non è coperto da borse di studio, mentre nelle altre Regioni del Paese il dato scende al di sotto del 10 per cento e, in alcune del Nord, anche al di sotto del 5 stiamo bruciando una generazione di ragazzi meridionali e non ne usciremo se non variamo - ecco dove sta la grande pecca del DEF 2016 e di questo Governo, che pervicacemente non vuole affrontare la questione meridionale specialmente

rispetto alle altre Regioni del Paese ed è una grave ipoteca per qualsiasi piano di riavvio delle Regioni meridionali. Fin quando nel DEF non ci sarà una politica per il Mezzogiorno basata sull'istruzione e l'alta formazione, il Documento non sarà votabile anche soltanto per questo argomento.

ancora una volta questo Governo continua ad apparire del tutto insufficiente. Il settore agricolo e agroalimentare occupa una parte assai piccola nel Documento in esame, pur essendo

Eppure il Governo non ne tiene conto. L'azione del Governo appare abbastanza insufficiente, perché non riesce a incidere ancora in maniera significativa. L'aumento continuo dei costi di produzione, la riduzione dei prezzi delle materie prime, le conseguenze del cambiamento climatico in atto, la concorrenza sleale, la contraffazione e l'aumento della tassazione sono ancora criticità di cui non volete tenere conto.

Continuate ad attuare misure di potenziamento che non sono a favore del settore agricolo e della pesca. Avete attuato una serie di stangate sul fronte fiscale, con l'aumento dell'aliquota della imposta di registro per i trasferimenti dei terreni agricoli (dal 12 al 15 per cento), con la rivalutazione dei redditi agrari, con l'aumento dell'IRPEF, oltre al sostanzioso taglio alla dotazione del fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli. Noi abbiamo proposto di introdurre misure di salvaguardia previdenziale e tutele sulle produzioni del comparto lattiero-caseario. Abbiamo tentato di disciplinare specifici

ma continuate a fare orecchie da mercante. Abbiamo proposto specifici interventi per rivalutare il settore anche in favore delle tecniche agronomiche, quali la permacultura. Un modo per poter aiutare il settore sarebbe stato offrire strumenti di sostegno alle filiere produttive con produzioni di elevata qualità garantire l'accesso al microcredito, che ancora aspettano le aziende dei settori della pesca professionale, del pescaturismo e dell'ittiturismo, proprio per dare una grande mano al comparto. Sempre nel settore della pesca, sarebbe stato utile operare nell'ambito delle competenze nazionali, per stabilire una disciplina chiara, trasparente e univoca in materia di distanze minime di pesca, non solo delle esigenze territoriali, ma anche della situazione morfologica del territorio, ferme restando, chiaramente, le norme sul fermo biologico e sulle esercitazioni militari. Abbiamo chiesto di attuare strumenti legislativi d'emergenza in favore degli imprenditori agricoli le cui attività ricadono in aree colpite da dissesto idrogeologico; introdurre adeguate misure per la semplificazione e la sburocratizzazione, per il riordino del sistema dei controlli, per la riduzione dei termini dei procedimenti amministrativi; di assicurare risorse aggiuntive alla legge n. 157 del 1992, in considerazione proprio dei continui danni agricoli provocati dalla fauna selvatica.

L'agricoltura e la pesca rappresentano la storia produttiva del nostro Paese, a cui devono essere restituiti i valori scippati dai vostri Governi degli ultimi anni; Governi fatti di braccia rubate all'agricoltura, che perseverano perseverano a derubare le ultime braccia rimaste e sopravvissute alle vostre cattive pratiche. Ci si augura solamente che il comparto agricolo risorga,

in analogia con quanto succede in altri Paesi, ma con un'intensità sicuramente riconosciuta da tutti (compresa la Corte dei conti) come la più elevata, sta cercando di recuperare tutti i margini di maggiore efficienza all'interno di questo settore. Siamo partiti da una spesa molto più bassa di quella di Francia e Germania e che garantiva risultati migliori rispetto a tali Paesi, ma stiamo intervenendo con restrizioni piuttosto consistenti da parecchi anni, che costringono le Regioni a riorganizzazioni molto pesanti. Nei limiti in cui si recuperano margini di efficienza, questo ovviamente non solo è dovuto, ma va sostenuto a tutti i livelli. Quello che ci preoccupa è il fatto che negli ultimissimi anni sempre più ci siano segnali di difficoltà difficoltà da parte dei cittadini ad accedere ai servizi. E non solo, ma sta anche emergendo dai dati ISTAT il timore da essi denunciato, che ormai credevamo superato, di non avere i soldi per curarsi di fronte a servizi sanitari che, sempre più,

la qualità dei servizi e l'equità di accesso ai cittadini. Con riguardo alle previsioni contenute nel DEF, la Commissione sanità ha fatto un'analisi molto puntuale, di cui sintetizzo soltanto gli aspetti più importanti. Intanto il dato della spesa 2015,

sanitario difficilmente riescano a portare a risultati concreti e finiscano per creare nel tempo l'accumularsi di situazioni di grande squilibrio fra entrate e spese.

la dotazione e la situazione del personale. Noi continuiamo ad avere in vigore una serie di tetti di spesa e di dotazioni che impongono una riduzione del personale dipendente. Questo rende difficile la situazione in un settore che produce servizi e che, quindi, confida nel principale fattore produttivo, che è il personale, tra l'altro sempre più anziano, sottoposto a turni sempre più elevati e soprattutto sempre più sostituito da forme di

- andrebbe gradualmente presa in considerazione, a partire dalla revisione dei contratti. Il secondo elemento riguarda i farmaci innovativi, che possono produrre risultati in termini di riduzione della mortalità o di situazioni gravi del

la mancanza, per ancora un altro anno o per più anni, di una ripresa degli investimenti in edilizia e in tecnologie sanitarie, che non soltanto consentirebbe di superare forme di obsolescenza e di vetustà ormai difficilmente

Signora Presidente, Vice Ministro, onorevoli colleghi e colleghe, il Documento di economia e finanza produce l'atto fondamentale per una pianificazione strategica politica ed economica a breve e medio periodo. Nel DEF 2016 sono le poche indicazioni e le altrettante poche certezze a emergere. Mancano informazioni dettagliate di misure alternative chiare e credibili al fine del consolidamento dei conti; insufficienti quindi per valutare se il programma di Governo possa essere credibile rispetto alla reale decrescita del debito. Manca una seria politica per un programma di investimenti a medio e lungo termine, che comporta molta incertezza, quella stessa incertezza che rallenta ulteriormente la ripresa tanto agognata. Lo stesso ISTAT, le cui valutazioni sono per natura asettiche, ha espresso perplessità, come peraltro lo stesso Ufficio parlamentare di bilancio, che vede il Paese esposto a importanti rischi. L'assenza di inflazione rappresenta il maggior rischio per l'andamento del debito, una variabile che non può essere sottovalutata. anche su alcuni obiettivi chiave, fondamentali per il fine ultimo, quale il rilancio della crescita e dell'occupazione, a partire dalla riduzione del debito, chiedendoci quanto possa essere credibile. Gli obiettivi legati agli incassi per le privatizzazioni sono forse troppo ambiziosi e, al momento, le conferme anche in questo caso sono insufficienti a fronte di un eccessivo ottimismo. Mancano indicazioni sulle alternative alla cessione di Ferrovie. le clausole di salvaguardia, non si comprende come saranno neutralizzate. Il paventato aumento dell'IVA creava una situazione di non chiarezza e una percezione di grande insicurezza. Vorremmo ora capire su quali partite si gioca il superamento.

e ponendo molti dubbi sui margini di risparmio dal lato delle spese, che potrebbero rivelarsi limitati per i prossimi anni. L'applicazione dei costi standard deve vedere un'accelerazione e necessita il superamento della spesa storica. Il controllo dell'evasione fiscale va legato a una minore pressione fiscale. È necessaria una riduzione delle tasse e va ripensato in modo strutturale l'intero sistema fiscale. Anche l'incertezza per le agevolazioni fiscali ha un peso determinante sugli investimenti e, quindi, sul rilancio dell'economia. Affermazioni quali una riduzione rilevante del tasso di disoccupazione non trovano riscontro nell'analisi attuale riferita al *jobs act*: crollo del 74 per cento per i contratti stabili, aumento dei *voucher* per le occupazioni occasionali. Ovviamente ciò crea incertezza per il futuro, specialmente tra i giovani che, purtroppo, fuggono all'estero. Parliamo di enti locali. L'abbandono del Patto di stabilità interna, che poteva dare respiro, ora con il pareggio di bilancio vede i Comuni in difficoltà, specialmente i piccoli, con i nuovi limiti imposti dall'autonomia finanziaria, non essere più in grado di sopportare i tagli: penso ai Comuni montani, ai Comuni della mia Provincia, del bellunese, che devono far fronte all'erogazione di servizi necessari e dovuti verso una popolazione sempre più anziana. minori le risorse per maggiori e più capillari servizi. Servono le necessarie risposte a famiglie e imprese per fermare lo spopolamento delle aree montane, le cui specificità sono riconosciute anche dalla legge n. 56 del 2014, meglio nota come legge Delrio, che le individua per quelle aree interamente montane confinanti con Paesi esteri. esteri. Chiedo per questo che il Governo dia le necessarie risorse, perché la parola "specificità" riassuma significato e dignità. l'ultimo rapporto del CER stima, per il primo trimestre del 2016, una crescita del PIL dello 0,8 per cento su base tendenziale e dello 0,2 per cento su base congiunturale. La crescita acquisita per l'intero anno risulterebbe pari a 0,5 punti. Ciò è a conferma del troppo ottimismo e della troppa incertezza espressi in questo DEF 2016 e ribadisce il nostro voto contrario, dovuto sicuramente a tutte le motivazioni espresse, le quali non danno né certezze, né sviluppo, né possibilità futura di avere per questo Paese una ripresa veloce necessaria

un Documento importante come il DEF meriterebbe maggiore attenzione da parte dell'Assemblea, perché in esso si guarda ai conti del passato e si progetta il futuro,

Limiterò il mio intervento all'esame di alcuni parametri che fotografano la drammatica condizione economica in cui versa il Paese. Il debito pubblico è ancora un problema, almeno fino a quando il costo non sarà pari a zero. sono previsti 67 miliardi per spesa, un po' meno degli 85 che abbiamo pagato in passato, ma si tratta sempre di risorse molto importanti.

le manovre finanziarie costate lacrime e sangue agli italiani. Ma è solo questo il dedito pubblico italiano? i 70 miliardi di debiti che la pubblica amministrazione ha nei confronti delle aziende, un dato in crescita piuttosto che in diminuzione; i debiti occultati dalle aziende sanitarie,

debiti dei Comuni, costretti addirittura ad aumentare la leva fiscale. Forse vi sfugge che ormai circa il 30 per cento dei cittadini non paga più l'IMU, la tassa sui rifiuti, la mensa, i trasporti ormai anche i Comuni sono destinati al fallimento, almeno tutti quelli che sono in seconda fila sulla costa, dove non ci sono le seconde case, le cui tasse ancora ne reggono le entrate. Ricordo

Ad ogni DEF avete annunciato il miglioramento di tale rapporto, che però puntualmente non si è mai realizzato. Questa volta prevedete un calo di tre decimi di punto, che sarebbe un miracolo,

come realizzeremo. E poi non prendiamoci in giro: pensare di ridurre il debito pubblico attraverso le privatizzazioni è - Non si possono vendere i gioielli di famiglia per tappare i buchi di bilancio.

Comprendo che le previsioni si debbano fare con una visione ottimistica (se si avesse una visione pessimistica, sarebbe anche peggio), ma non bisogna esagerare. Le previsioni contenute nel DEF del settembre 2013

Credo che la vostra previsione di crescita non si realizzerà. L'avete collocata nella forbice verso il limite massimo, ma ritengo che un buon Governo debba essere cauto e prudente. Voi siete troppo ottimisti, perché siamo di fronte a un quadro economico internazionale di grande incertezza in virtù di una grande debolezza della ripresa globale.

Non va meglio nel campo della produzione, dove si assiste alle smantellamento del settore che una volta era secondo in Europa solo a quello della Germania.

L'Italia si colloca ai primi posti tra le maggiori economie europee per il peso del cuneo fiscale. Nel 2015, secondo l'OCSE, la pressione tributaria e contributiva su un capofamiglia con due bambini è stata pari al 39,9 per cento del

di conseguenza la pressione fiscale, perché voi prevedete 5 miliardi di aumento di entrate, da 784 a 789 miliardi di euro nel 2016,

Sempre più anziani non hanno i soldi per curarsi. La salute è andata a farsi benedire. Per la prima volta in Italia l'aspettativa di vita è in calo (-0,2, -0,3 dai tagli nei servizi sociali. I fondi per le spese sanitarie scarseggiano e nel DEF sono previste ulteriori riduzioni. Nei primi mesi dell'anno - questo è veramente drammatico i decessi sono stati 445.000 contro i 399.000 dello stesso periodo dello scorso anno, un'impennata dell'11 i morti saranno 166.000, livello mai toccato in Italia dal 1945.

Hanno peggiorato negli ultimi anni il livello di alimentazione; sono stati costretti a dormire per strada; chi cammina per Roma vede quante persone dormono per strada e com'è cambiata la situazione rispetto al passato. la crisi si sta riversando sempre più sulle spalle delle fasce più deboli. Noi crediamo che le vostre politiche economiche siano inadeguate e sbagliate nonostante condizioni congiunturali siano molto favorevoli. Il costo del denaro si è ridotto di molto ed è passato dal 5,2 al 4,2 per

gli ultimi dati resi noti ieri rappresentano un preoccupante e netto calo delle esportazioni verso i Paesi extraeuropei del 5,2 per cento su base annua. la vostra esultanza, rappresentata dal Presidente del Consiglio una settimana fa qui, è del tutto fuori luogo. Siamo di fronte ad un aumento del debito pubblico, alla chiusura di aziende e all'aumento della disoccupazione. In sostanza, i vostri conti sono sballati. Avete poca credibilità nelle vostre previsioni. Il Paese sta andando verso il baratro.

ci dava il quadro della pesantezza della crisi che abbiamo vissuto nel mondo, in Europa e nel nostro Paese.

inferiore di quattro punti rispetto alla media europea. Ciò significa che abbiamo perso 21 punti di PIL *pro capite* rispetto alla media europea. Dopo Grecia e Cipro siamo il Paese più colpito dalla crisi negli anni fatidici della recessione del 2007 e del 2008, con una riduzione del prodotto interno lordo di 10 punti. un dato ben peggiore di quello della crisi del 1929 per quanto riguarda il nostro Paese, con un calo dei consumi dell'otto

non abbiamo avuto ulteriori decrementi del prodotto interno lordo: 2,8 per cento nel 2012, 1,7 nel 2013, 0,3 nel 2014.

senza responsabilità politica. Vorrei ricordare all'ultimo collega intervenuto, che accusava il Governo di non fare nulla, di sbagliare la ricetta, che la crisi di quegli anni Fu un Governo di centrodestra, presieduto dal presidente Berlusconi, a portare il Paese in quella condizione. In questi anni abbiamo cercato di scalare una montagna per ripartire da quella situazione in una fase in cui non siamo all'interno di una congiuntura economicamente positiva a livello internazionale ed europeo; anzi, la situazione in Europa ci vede contrapposti alle ricette di austerità (contro la flessibilità) che vengono portate avanti

Banca centrale tedesca, che ancora oggi continua a portare avanti l'idea di politiche di austerità come unica possibilità per risanare il bilancio e far ripartire l'economia. Ecco, da questa situazione siamo ripartiti, con questo livello di contrasto e di difficoltà, e però oggi possiamo dire che il Paese è uscito dal *tunnel* perché in questo Documento leggiamo che nel 2015 abbiamo avuto un risultato dello cento di crescita del prodotto interno lordo. Per la prima volta abbiamo un dato consolidato che inverte la tendenza: abbiamo un segno

sforamento è solo dello 0,1 per cento. Quindi, i dati che il Governo inserisce nel DEF non sono contestabili, messi da chi vuole dipingere

dell'occupazione. La disoccupazione si è ridotta di 0,8 punti percentuali, attestandosi oggi all'11,9 per cento. Certo, non è ancora sufficiente, dobbiamo andare avanti, ma anche in questo caso, per la prima volta, c'è un segno positivo dovuto alle politiche del Governo, alle riforme

C'è stata una ripresa degli investimenti, una ripresa consistente dei consumi. Oggi siamo un Paese che cresce

ci siamo divisi ed abbiamo discusso; però non possiamo negare e nessuno di noi può contestare il fatto che oggi siamo passati da una fase in cui discutevamo delle riforme ad una fase in cui le riforme le approviamo e le facciamo. Per questo oggi abbiamo una considerazione diversa in Europa e per questo oggi il nostro Presidente del Consiglio - e vorrei che

per l'Europa una politica diversa, non più di austerità e con margini maggiori di flessibilità, che sono anche all'interno di questo Documento di economia e finanzia. Credo che siamo sulla strada giusta e che il Paese stia capendo che, per la prima volta, ce la possiamo fare. Signor Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi senatori, non mi eserciterò nell'inutile tentativo di individuare responsabilità e colpe e di dare letture addomesticate o addomesticabili dei numeri relativi alla condizione del Paese. Certo, vorrei che fossero tutte inconfutabilmente

di cui egli parla e di cui, a mio avviso, purtroppo il nostro Paese non gode, né in Europa, né nel mondo, se è vero, com'è vero, che siamo vittime della prepotenza di

dei marò restano irrimediabilmente pagine nere, che mortificano il tricolore e che certamente non indicano un livello di credibilità internazionale che pure desidereremmo fosse rilanciato. La verità è che in abbiamo 1.300.000 minori che vivono in una condizione di grave deprivazione e di perdurante disagio. L'11,5 per cento delle famiglie affonda in uno stato di povertà assoluta. Le aziende arrancano e continuano a chiudere, sotto i colpi di una tassazione che non ha pari in Europa. che considero allarmante e che non sono il solo - come dirò fra poco - a considerare tale, c'è un caso Sud che è sempre più in fondo a tutte le classifiche di crescita, ma primo purtroppo in tutte quelle relative alla disoccupazione, al disagio sociale e all'inadeguatezza strutturale, tagliato fuori dall'agenda del Governo,

la finalità e l'esito della lettera che, proprio ieri, il Presidente della Regione Puglia ha inviato al Primo Ministro per sapere se, come e quando verranno destinate le risorse dei fondi per il Mezzogiorno

La crescita è abbarbicata intorno allo "zero virgola". Il 10 per cento delle famiglie addirittura rinunzia a curarsi e, per la prima volta negli ultimi dieci anni, si riduce perfino l'aspettativa di vita degli italiani. A dircelo è proprio il rapporto presentato ieri da Osservasalute, che individua la causa di questa riduzione delle aspettative di vita

a scattare la fotografia puntuale e precisa. L'impresa ci dice che nei prossimi quattro anni le uscite dalle casse dello Stato cresceranno sempre di più, con un incremento complessivo di 22 miliardi di euro, la spesa pubblica

Tra il 2016 ed il 2019, una stangata fiscale da oltre 71 miliardi di euro. Aumenteranno sia le imposte dirette sia le imposte indirette: nel primo caso il Governo

nei prossimi quattro anni le tasse rischiano di aumentare progressivamente ogni anno e il gettito complessivo supererà la quota di 855 miliardi di euro rispetto ai 785 miliardi

disegnano un quadro che - purtroppo - rappresenta ancora l'identità di un Paese che versa in una condizione di difficoltà gravissima. Sono dati che non si possono confutare. Metto in fila questi numeri perché niente al pari dei numeri può dimostrare la fragilità e la precarietà del Documento di economia e finanza in esame, cogliendo di fatto in fallo il Governo che tenta - così pare - di raccontare un'altra verità. Governo ci racconta di un Paese che è uscito dalla stagnazione economica per un solo «zero virgola» con il segno «più» e in cui le aziende hanno ripreso a investire,

Primo Ministro relative al fatto che le famiglie italiane si sono arricchite. Un Paese dove le persone che vivono dentro l'area del disagio e della povertà stanno diminuendo e dove nessuno più si toglie la vita quando la disperazione, purtroppo, ha il sopravvento sulla speranza. Noi vorremmo davvero che fosse così, ma quel senso di disperazione, angoscia e inquietudine purtroppo serpeggia ancora nel Paese. Non si tratta solo di una questione di ottimismo o pessimismo relativo ai titoli dei giornali e a a quel che si dice nei *talk show* televisivi: è la situazione di sofferenza scritta nella storia quotidiana di gente che non ce la fa più. L'Ufficio parlamentare di bilancio, la Banca d'Italia, l'ISTAT e la Corte dei conti raccontano un'Italia diversa da quella che si legge nel DEF e nelle parole di rassicurazione che di recente, anche in quest'Aula, abbiamo sentito dal Presidente del Consiglio. In occasione delle audizioni

a sottolineare come la lentezza anomala con cui cresce l'Italia determinerebbe un'esposizione al rischio, con particolare riferimento alla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia che, seppure condivisibile, genera - viene detto - nei fatti ambiguità e incertezza, perché non è supportata da una credibile politica di riforme, di taglio della spesa pubblica improduttiva e di contestuali misure per contenere i conti. il Documento in esame rischia di essere privo dei necessari caratteri di attendibilità e credibilità nella prospettazione delle linee di politica economico-finanziaria. Manca un atteggiamento prudente da parte del Governo. Le indicazioni contenute nel DEF sono aleatorie, tanto più di fronte alle recenti affermazioni del Presidente del Consiglio, rese anche in quest'Aula, in merito alla volontà di procedere a un abbassamento della pressione fiscale: un obiettivo necessario, necessario, condivisibile, da sostenere, ma realizzabile con altro tipo di presupposti e con differenti condizioni. Noi, come Gruppo dei Conservatori e Riformisti, abbiamo invocato da tempo questa strada, ma abbiamo nel contempo indicato, anche attraverso l'attività emendativa, la strada delle relative, indispensabili coperture di spesa perché il taglio fosse possibile. Invece, in questo caso, il taglio delle tasse è evocato senza fornire delucidazioni persuasive. È la Corte dei conti, in particolare, a sottolineare come per tagliare le tasse - cosa necessaria e non più rinviabile - occorra mettere mano a una riforma strutturale del sistema tributario; riforme strutturali che il Governo fa finta di fare, quando le fa, aiutato anche da una maggioranza che spesso dissente fuori da quest'Aula, ma che poi, nei fatti, vi acconsente al suo attraverso il supporto a provvedimenti che hanno assolutamente dubbia se non scarsa efficacia, a iniziare da quelli sulla scuola, per proseguire con le politiche del lavoro e delle pensioni. La stessa Corte dei conti suggerisce il percorso per tagliare le tasse: l'ampliamento della base imponibile, la rivisitazione degli obiettivi redistributivi assegnati ai sistemi di prelievo, la ricerca di un effettivo coordinamento della leva fiscale tra livelli di Governo. assistiamo a un sistematico scaricabarile tra Governo, Regioni e Comuni che produce l'effetto *boomerang*. Ne è la riprova

La pressione fiscale è rimasta, così, superiore per 2,5 punti percentuali alla media registrata nel decennio precedente alla crisi dei debiti sovrani. Un discorso a parte merita la sanità. Siamo di fronte a un Documento che lascia irrisolte alcune criticità importanti sul piano della sostenibilità del sistema sanitario, unitamente alla necessità di mantenere l'equilibrio tra garanzie ai cittadini e organizzazione dell'offerta, con l'obiettivo di rendere la spesa pubblica per la sanità sostenibile senza pregiudicare la qualità dei servizi e l'equità di accesso alle cure. Non solo: vengono amplificate le contraddizioni, che sostanzialmente inseriscono voci come le risorse umane in una fantomatica *spending review*, anziché porle tra le voci di investimento e, giocando tra spesa e finanziamenti, si lasciano impregiudicati gli sprechi, mentre i livelli essenziali di assistenza si abbassano e in alcune Regioni sono addirittura pregiudicati, rispondendo a logiche che riducono la sanità a un puro e semplice aggregato di beni

Quando si parla di beni così delicati bisogna recuperare il principio di responsabilità, imparando in Aula e nelle sedi istituzionali la lingua della verità. Attraverso l'analisi corretta della difficile situazione economica

la riconnetta al Paese, in una logica virtuosa e di recupero della credibilità, ma che sia capace anche di disegnare una prospettiva destinata al recupero della fiducia e della speranza. Questa è un'occasione perduta perduta per dire agli italiani la verità e per dare loro una prospettiva di sviluppo seria e credibile, costruita con senso di responsabilità. Prevalgono invece la consapevole sottovalutazione

la questione delle infrastrutture di rete e la banda larga. Il Governo aveva approvato il programma operativo del piano per la banda ultralarga, ed erano stati assegnati 2,2 miliardi di euro a valere sul Fondo sviluppo e coesione. Ci sembrava un passo importante per un Paese come il nostro

cercando di far capire con diverse azioni che potremmo trovarci con un grosso problema in un futuro non troppo lontano. Ci sono importanti e ingenti risorse che possono essere messe a disposizione, ma ci sono troppe questioni alle quali il Governo non riesce a dare risposta; e questo viene anche sollecitato da parte degli operatori. Noi corriamo un rischio perché il Governo non fa il regista, non esercita il suo ruolo attraverso il comitato per la diffusione della banda larga, che dovrebbe vigilare su questa importante operazione; regna la confusione e gli operatori non sono contenti; manca il catasto delle reti. Noi vogliamo mettere fibra ottica nel Paese, ma non sappiamo quanta fibra ottica c'è, quanta di questa - come viene detto tecnicamente - è spenta (perché la verità è questa) e come si fa progettare una rete nel Paese quando non si sa cosa abbiamo sotto i piedi. Manca la regia.

fermo al neolitico per quanto riguarda il sistema della banda larga. Oltre ad avere un *gap* generazionale all'interno della nostra società, stiamo pagando pesantemente scelte fatte in maniera inconsueta rispetto ai nostri *partner* europei da parte di Telecom, che purtroppo scontiamo ancora oggi.

di ritrovarci tra qualche anno con addirittura due reti sovrapposte, ancora una *incumbent* come la avevamo prima, che non creerà quella rete che noi speriamo tanto di avere, ossia una rete libera con la parità di accesso da parte di tutti gli operatori. Staremo a vedere, come abbiamo detto più volte. Veniamo al secondo punto, quello delle opere pubbliche e delle infrastrutture. Devo dire innanzitutto una cosa al vice Ministro; ha vinto la linea Padoan,

ci lascia molto perplessi e ci lascia l'amaro in bocca, perché l'anno scorso avevamo chiesto al Ministro che oltre alle famose 25 opere, le uniche

per gli investimenti in materia di trasporti non si prevede la lavorazione di un nuovo allegato infrastrutture al DEF. Ciò per una ragione molto semplice; è la strategia di Renzi. Non si scrivono nomi e cognomi delle opere, in modo che potrà poi scegliere in maniera discrezionale. Renzi potrà gestire in maniera discrezionale le opere, però - guarda caso - e lo diciamo ancora oggi, così resterà agli atti, nelle 25 opere abbiamo trovato ancora una volta la tramvia di Firenze. Tale tramvia è sicuramente strategica nel quadro generale delle grandi opere infrastrutturali del Paese. Ho anche cercato, signor Vice Ministro (ma non sono riuscito a trovarla), tra le 25 opere quella forse più importante,

fra i circa 40 milioni di elettori qualcuno pensa che abbiamo dato lezioni anche a quelli che sono maestri a fare infrastrutture in Europa. Questa è la strategia di Renzi: raccontare un sacco di balle. raccontare un sacco di balle. Siamo arrivati al punto di essere così spudorati. Speravo veramente che con il ministro Delrio, che più volte in Commissione è venuto è venuto con tutte le buone intenzioni, dicendo che addirittura aveva parlato della cura del ferro per le infrastrutture del Paese, ci fosse davvero un cambio di passo. Volevamo davvero avere una lista di opere serie da fare in questo Paese, cancellando quelle che erano descritte - e qui siamo d'accordo

la cosa finirà nel ridicolo. Vi siete riempiti la bocca anche sulla questione della riforma del codice degli appalti, dicendo che sarà una rivoluzione. Sì, una rivoluzione per morire nel ridicolo, perché perché sempre all'interno della discrezionalità le opere andranno ad insabbiarsi perché avete inserito, in maniera molto maldestra, la questione del dibattito pubblico per quanto riguarda le infrastrutture, in maniera talmente bizantina e distorta che andrà ad insabbiare le opere pubbliche. Questa è una scelta che sicuramente dà una mano alla volontà di questo Governo di voler fare le opere con discrezionalità, con discrezionalità, senza programmazione sul territorio, con una visione assolutamente miope, mai vista in questo Paese che già non brilla per quanto riguarda le opere pubbliche. Ricordo sempre, però, che ci sono Regioni e Province

Signor Presidente, colleghi, in questo anno molti nodi stanno venendo al pettine e non ci sarà nessun piano Juncker a salvarci. Invocando l'Unione europea vogliono toglierci risparmi, diritti e democrazia. L'Unione europea in costruzione ci sta inesorabilmente impoverendo, incurante dell'esistenza delle nostre microimprese, refrattaria a riconoscere le nostre tipicità, ma pronta a bacchettarci non appena si accorge che non abbiamo fatto i compiti a casa. Un'Unione europea nella quale noi italiani abbiamo un membro del Governo che, evidentemente, invece di tutelare i nostri interessi, sembra essere troppo prono ai voleri di Bruxelles, nonostante ci siano molti esempi di come gli Stati membri, spesso, disattendano le decisioni della Commissione europea. In qualche misura il DEF e la politica economica ad esso sottesa rappresentano bene la posizione del Governo: aspettiamo la crescita, poi vediamo cosa fare. I provvedimenti a favore delle aziende sono stati realizzati: il mercato e le imprese sanno cosa fare. Qualora si aprissero nuovi spazi finanziari, per esempio una contrazione dei tassi di interesse relativi al servizio del debito pubblico, è possibile prefigurare delle misure procicliche. Il DEF riduce la politica pubblica a semplice cornice dei fenomeni. Al Governo sono convinti che la crescita economica arriverà, occorre pazienza. Appena la crescita si manifesterà, tutte le operazioni di finanza pubblica diventeranno plausibili e politicamente sostenibili. Secondo il *Premier* e Ministro dello sviluppo economico, le tasse sono diminuite e continueranno a farlo. L'atteggiamento è quello tipico delle politiche neo-liberiste: solo la riduzione delle tasse può far crescere l'economia, con un atto di fede e di fiducia nel mercato e nelle imprese spropositato. Se poi non dovesse realizzarsi la crescita, vuol dire che si sono ridotte le tasse troppo poco o che non si è flessibilizzato abbastanza il mercato del lavoro. Peccato. Nel frattempo sono intervenuti il *quantitative easing* di Draghi e il calo del prezzo del petrolio al barile. Se la riduzione del costo del lavoro italiano è prossima a quella dei Paesi periferici dell'Unione europea, il contributo modesto delle esportazioni alla crescita del PIL nasconde qualcosa di più preoccupante. Ciò che il Governo nasconde accuratamente è la distanza dell'Italia rispetto alla crescita media europea, che nel corso degli anni si è consolidata e poi ampliata. Se il *quantitative easing* e il deprezzamento del petrolio sono positivi per la crescita (sempre che sia vero in assoluto), una riduzione del prezzo del petrolio potrebbe avere anche un effetto negativo sulla domanda dei Paesi che lo esportano e sullo sviluppo delle tecnologie rinnovabili è altrettanto vero che i benefici sono orizzontali e valgono per tutti i Paesi. Forse un problema di struttura il Paese lo deve realmente affrontare, diversamente dalle riforme strutturali che intervengono sempre a margine di un dato sistema produttivo. La difficoltà dell'Italia nell'agganciare la crescita economica nella misura degli altri Paesi consegna alle riforme strutturali un peso-valore in verità Dal lato occupazionale non si vedono grandi scostamenti: solo i consumi e gli investimenti segnano un miglioramento che mal si concilia, però, con l'andamento della stessa occupazione. Come può aumentare il consumo se il tasso di occupazione rimane stabilmente al di sotto della media europea? Evidentemente qualcosa non funziona nel modello utilizzato: o le riforme fanno crescere il PIL e quindi migliorano i conti pubblici, oppure la crescita del PIL è incerta. tuttavia, è quella dei tagli di spesa pubblica o la conseguente clausola di salvaguardia, che riducono la domanda aggregata e quindi il PIL. In realtà, lo scopo dell'unità monetaria europea (quindi, a cascata, delle politiche economiche dei Paesi dell'eurozona) è quello di trasferire sul mercato del lavoro il normale aggiustamento degli *shock* esterni, che abitualmente nel resto del mondo si verifica attraverso l'aggiustamento del tasso di cambio. Pertanto l'Unione europea e l'eurozona, non potendo cedere il valore della moneta, hanno ceduto il valore dei salari e, quindi, i Paesi europei del Sud sono entrati in deflazione. Il Governo ha svenduto molti gioielli italiani con scarsissimi profitti; nemmeno Amato nel 1992 aveva fatto tanto e sappiamo come è andata a finire, ma allora almeno era ben definita una politica industriale, seppur scarsamente condivisibile. Pensare di ridurre il debito privatizzando è ormai una menzogna consolidata. Ormai sono chiare le intenzioni di questa politica economica: le logiche di mercato devono sostituire lo Stato sociale e le Costituzioni, determinando la compressione dei redditi da lavoro degli Stati europei.

e credo che sia sensato fare un breve riepilogo dello stato dell'arte, il vice ministro Morando certamente conosce e ha l'incombenza di dover affrontare. La dichiarazione è icastica: noi siamo un Paese in braghe di tela. Siamo un Paese nel quale le prime quattro voci di spesa, che assorbono quasi tutto quello che riusciamo a spendere, sono rappresentate dalle pensioni, dagli stipendi ai 3,5 milioni di impiegati dello Stato, per 111 miliardi di euro dalla sanità e per 80 miliardi di euro dagli interessi passivi sui 2.200 miliardi di euro di debito. Questi sono i limiti e gli ambiti all'interno dei quali il Governo, qualunque Governo, deve muoversi. senza questa considerazione sull'effettiva consistenza economico-finanziaria dello Stato ogni critica diventa artificiosa, così come ogni plauso diventa una

facendo piccoli aggiustamenti sui vari capitoli di spesa, non certo ottenendo dall'Unione europea maggiore flessibilità, ma convincendoci tutti quanti, tutti coloro che hanno responsabilità nelle varie istituzioni del Paese, che la Nazione ha bisogno di profonde riforme dell'organizzazione, della funzione e dei compiti assegnati allo Stato. Finora abbiamo avuto un Governo che si è timidamente affacciato alla stagione del riformismo, ovviamente tenendo ben presente che ha ereditato cinquant'anni di gestione dello Stato attraverso la leva della spesa e del debito crescente. È quindi una politica che oserei definire keynesiana - se mi si consente il termine - nella quale lo Stato diventa di per se stesso chi ci accompagna dalla culla alla bara. Lo Stato diventa di per se stesso il più grande capitalista in questa Nazione con le sue circa 10.000 partecipate

partecipate dallo Stato? Quando faremo, in via definitiva e irreversibile, la svolta liberale nelle istituzioni e daremo al libero mercato di concorrenza la possibilità di permeare non solo l'economia, ma anche tutti gli ambiti d'intervento dello Stato? Stato? Dico questo perché, se alle precedenti generazioni di dirigenti dello Stato è stato facile e comodo riconoscere diritti e accontentare i contemporanei (che votano e protestano) per addebitarne il costo ai posteri (che non votano e non protestano), questo non ci è più consentito. Non ce lo consentono l'Europa, i rigidi vincoli che l'Unione europea ha posto sulle spalle dell'Italia; non ce lo consentono i 2.200 miliardi di euro di debito.

della produttività, dell'efficienza e del rapporto costi/benefici. È chiaro che, poiché i clienti di mestiere fanno gli elettori, questo non può che portare ad uno scadimento del consenso nei confronti del Governo. Poiché viviamo l'epoca dello sciacallaggio politico e dell'odio in servizio permanente ed effettivo, perdiamo tempo appresso alle tesi moralisteggianti e strampalate di quelli che pensano che uno Stato in queste condizioni si possa salvare al grido di «onestà, onestà», quasi che l'onestà, di per se stessa, facesse grazia a chi governa un Paese di 60 milioni di persone del dovere di avere la capacità di scegliere tra modelli di Stato che sono alternativi. Lo Stato socialista muore di socialismo; lo Stato socialista muore di partecipazione dello Stato, di monopoli, di disservizi e anche di corruttela.

perché il libero mercato si svolge all'interno di regole. Quando chiesero a Karl Popper quando si sarebbe applicato il liberalismo nell'Unione sovietica appena caduto il Muro di Berlino, sovietica appena caduto il Muro di Berlino, egli rispose: lo applicheremo non appena avremo uno Stato e istituzioni in grado di dare regole e leggi a questo Stato all'interno del quale la competizione possa avvenire. Signor Vice Ministro, la mia benevola astensione dal giudizio perché lei gestisce quello che ha ereditato. Quindi, noi la giudicheremo più sulle prospettive

Credo valga la pena citare soprattutto tre dati: è diminuito il costo del lavoro, è aumentata l'occupazione e il Paese è in crescita con un saldo positivo dello 0,8 La crescita è merito del coraggio di tanti imprenditori, della voglia degli italiani di rimboccarsi le maniche e lasciarsi alle spalle gli anni duri della crisi, ma è anche merito del Governo e del Parlamento, che hanno saputo dare attuazione, come ci viene ricordato da una puntuale analisi pubblicata su «Il Sole 24 Ore», a più della metà della riforme che in questo tempo sono state approvate. Di questo va dato atto all'Esecutivo e alla maggioranza. Oggi l'Italia sembra essersi lasciata finalmente alle spalle gli anni peggiori di una durissima crisi che - non dimentichiamolo - ha riguardato tutto il mondo occidentale (per trovare precedenti bisogna risalire ai tempi della Grande depressione del 1929). Certo, lo 0,8 per cento di crescita è solo il timido inizio di un percorso ancora lungo per fare in modo che gli italiani sentano che il peggio è alle spalle, che il futuro non è una minaccia ma può tornare ad essere un'opportunità. In questo senso ho apprezzato le parole e il coraggio che il Presidente del Consiglio ha più volte speso a riguardo, non ultimo durante l'esame della mozione di sfiducia qui in Senato la scorsa settimana. Concordo con lui che questa debba essere la stagione del coraggio e della responsabilità. Mi appare un atto di grande responsabilità nei confronti del Paese l'atteggiamento prudenziale del Governo sia sui numeri contenuti nel DEF sia sul fatto che quelle che vengono indicate come leve principali della crescita - parlo della ripresa dei consumi interni e dell'aumento dell'*export* delle nostre aziende - potrebbero da sole non farcela a raggiungere l'obiettivo previsto (+1,2 per cento). Tutto questo suggerisce lo schema di lavoro dei prossimi mesi. Il DEF, non a caso, indica come prioritari due macrotipologie di interventi: nuovi investimenti di carattere pubblico e la riduzione del carico fiscale sulle famiglie e le imprese. Ne aggiungo una terza: politiche che incentivino il tessuto imprenditoriale a puntare sull'innovazione, sulla ricerca, sulla qualità e sulla promozione dei nostri prodotti. Solo in questo modo potremo aumentare il peso del *made in Italy* sui mercati internazionali e, allo stesso tempo, spingere le aziende ad investire, favorendo così anche la leva del consumo interno. Al riguardo, uno dei grandi nodi da sciogliere è quello della semplificazione burocratica, perché la burocrazia continua ad essere, per moltissime aziende, soprattutto le piccole, una vera e propria tassa occulta o comunque un freno per un pieno sviluppo delle loro potenzialità, oltre che, naturalmente, un altissimo costo per le casse pubbliche. Su questo tema, che è uno degli appunti mossi dall'Unione europea al nostro Paese, sugli obiettivi in merito alla semplificazione burocratica del DEF, credo che lo sforzo debba essere molto maggiore, affinché gli effetti positivi, in termini di PIL, siano raggiunti ben prima del 2020 per quel che riguarda lo 0,4 cento nel 2030. Bisogna fare prima, con più coraggio, con più forza. Contestualmente, occorre puntare su quelle misure che sono in grado di costruire circuiti virtuosi, da cui tutti gli attori in gioco - dal cittadino-consumatore, alle imprese, all'erario - ne traggono beneficio. Solo per fare un esempio molto concreto, ritengo significativo che quest'Assemblea abbia approvato, con il benestare del Governo, mozioni che chiedono di stabilizzare, per i prossimi tre anni, gli incentivi fiscali sugli ecobonus. Si tratta di una misura che, dati alla mano, ha prodotto importanti risultati anche sul terreno di un maggiore gettito fiscale. Io ed altri colleghi abbiamo chiesto anche altre misure e mi auguro che il confronto annunciato possa produrre misure sostanziose. Dobbiamo puntare di più sugli investimenti, sul credito alle imprese che vogliono crescere, sulle garanzie bancarie; oggi, purtroppo, il sistema non aiuta le imprese che vogliono investire. Le risorse impiegate sugli investimenti producono reddito, favoriscono i consumi e aumentano il gettito fiscale. In questo senso, salutiamo positivamente anche la menzione che il DEF fa al collegato sul lavoro autonomo e al provvedimento, adesso all'esame della Commissione finanze della Camera, per la riforma del sistema

In sostanza, credo che gli investimenti pubblici e la riduzione della pressione fiscale indicata dal Governo debbano essere inseriti in un ragionamento complessivo, con una sua coerenza interna, con una logica di indirizzo politico; altrimenti il rischio, come più volte è stato dimostrato in passato, è che queste misure si disperdano senza Solo per fare un esempio, mercoledì scorso una delegazione dell'Intergruppo parlamentare per lo sviluppo della montagna e dell'UNCEM ha avuto un incontro con il presidente Mattarella, che ha mostrato sensibilità e attenzione per la situazione delicata in cui versano i territori montani e le loro imprese e per le difficoltà che derivano da una burocrazia tarata per le imprese di pianura, che non tiene conto delle specificità di un territorio dove le imprese commerciali, per poter sopravvivere e garantire servizi essenziali, devono poter puntare sulla multifunzionalità o dove, ad esempio, gli agricoltori *part-time* devono essere tutelati, perché scongiurano l'incuria di un territorio che gioca un ruolo fondamentale contro il dissesto idrogeologico. Su questo ancora troppo poco è stato fatto e non mi stancherò mai di chiedere il più volte promesso collegato sulla montagna. Sui dati macroeconomici riportati nel DEF, ad iniziare da quelli sul debito e sul percorso di avvicinamento al pareggio di bilancio, da un lato non possiamo che riscontrare come l'Italia, in questi anni, abbia operato per rispondere alle attese dell'Europa, ai cui occhi siamo un Paese finalmente stabile e finalmente affidabile. Ma è anche vero che non è più tempo di politiche dell'austerità.

che apra spazi effettivi per una riduzione del carico fiscale e che possa essere davvero percepita come tale dai cittadini. È questo il vero punto dirimente. È importante la decisione europea di ridurre la flessibilità delle clausole sulle riforme e sugli investimenti; meno comprensibile limitarne l'effetto cumulato allo 0,75 per cento del PIL, così come il fatto che l'ambito delle circostanze eccezionali non includa i costi sostenuti per la sicurezza, per l'emergenza migratoria e per la lotta al terrorismo. Ritengo positiva invece un'altra iniziativa, appena intrapresa anche dall'Italia, per introdurre il graduale passaggio dal *deficit* strutturale all'evoluzione delle spesa pubblica, con lo scopo di rendere il Patto di stabilità più efficace, ma anche più trasparente agli occhi dell'opinione pubblica europea. Il punto vero è che ancora oggi non si riscontra, a livello europeo, quel cambio di passo necessario per abbandonare la stagione dell'austerità. Vi sono segnali ancora troppo timidi, a fronte anche delle incertezze legate all'andamento del prezzo del petrolio e al tasso di cambio dell'euro.

il nostro tessuto economico potrà assurgere pienamente alla funzione cui questo DEF in qualche modo lo chiama. Adesso però è il momento di spingere sull'acceleratore, proprio in virtù delle turbolenze e delle incognite che si vedono all'orizzonte. Tra queste, non possiamo assolutamente sottovalutare quello che sta succedendo al Brennero con la chiusura delle frontiere sia per i suoi risvolti economici, che per quelli simbolici, il cui portato è devastante. C'è, da parte mia e del nostro Gruppo, il pieno riconoscimento per quello che finora è stato fatto da questo Governo. In una situazione interna, europea e internazionale non affatto facile, il Paese è stato rimesso sui giusti binari; non era un fatto scontato e di questo ne va dato assolutamente atto. Ancora una volta siamo davanti a un passaggio decisivo e occorre fare il massimo possibile. Io credo che non ci sia altra strada. Presidente, ritengo che sia mio preciso dovere affrontare questa discussione e fare questo intervento con un'ottica mirata su uno dei temi che ritengo abbia un valore rispetto alle necessarie iniziative che devono essere poste in essere. non riguardano solo l'attività del Governo, ma riguardano l'attività più complessiva del sistema istituzionale, politico, economico e sociale di questo Paese,

decisivo per il Paese e per la sua capacità di produrre e costruire elementi e prospettive di sviluppo stabile superare questa divergenza tra un Centro-Nord che va a una certa velocità e un Mezzogiorno e le isole che, invece, patiscono tante difficoltà.

Nelle stesse cartine troviamo situazioni dove i tassi di disoccupazione sono fisiologici e raffigurano il tempo necessario per cambiare lavoro (ma il lavoro c'è sempre),

Ci abbiamo provato anche nel corso della discussione sull'ultima manovra finanziaria, dicendo che il problema del Mezzogiorno è centrale e che dobbiamo fare un'operazione di riequilibro territoriale.

di intervenire su processi di deindustrializzazione selvaggia e di smantellamento complessivo dell'apparato produttivo, di recuperare il valore dello sviluppo locale e di valorizzare le risorse (che pure ci sono nel Mezzogiorno d'Italia e che vanno messe a frutto). Essa riguarda altresì le vocazioni produttive di una parte d'Italia

ce li abbiamo tutti: abbiamo tutti i teatri dell'inquinamento ambientale, da quello militare (presente nei poligoni), a quello edilizio (dovuto all'intensità delle costruzioni soprattutto sulle coste), a quello di cave e miniere, a quello relativo all'attività industriale, soprattutto siderurgica (che ha lasciato tanti strascichi e che oggi è sostanzialmente abbandonata e chiusa, con vertenze aziendali che si protraggono costantemente). Concludo, signor Presidente, dicendo che noi presenteremo una proposta su questo tema, che non apre alcuna polemica con il Governo, ma che lo invita ad affrontare questo argomento con un piano organico di interventi che sappia che sappia modificare lo stato delle cose a favore di quelle comunità, di quei territori e di quelle popolazioni. Signor Presidente, basterebbero dieci secondi, in sintesi, per illustrare la dinamica del DEF: crescita del PIL 2016 rivista al ribasso; rapporto debito-PIL che cala meno del previsto; ufficializzazione - anche se tra le righe - della necessità di un aggiustamento di quasi 2 miliardi dei conti pubblici; richiesta all'Unione europea di altra flessibilità, per la bellezza di 11 miliardi di euro, anche per il 2017. Renzi nel DEF riduce le stime di crescita economica per il triennio 2016-2018 e rivede l'aumento del PIL reale, che scende all'1,2 per cento rispetto allo sbandierato 1,6 Lo scenario economico, in pratica, si fa via via più fragile. Di fatto, l'Italia chiede all'Europa di poter aumentare il *deficit* di 11 miliardi rispetto al previsto. Il Governo passa in rassegna le politiche di sostegno alle imprese, dalle misure che afferiscono all'accesso al credito, a quelle relative al sostegno agli investimenti tramite sgravi fiscali e incentivi dedicati. Per rendere più competitive le imprese italiane è essenziale stimolare la spesa in ricerca e innovazione. Di fatto, il Governo non indica interventi specifici di potenziamento, né velocizza interventi già previsti, come nel caso del Programma nazionale della ricerca. Non si evincono interventi migliorativi per potenziare l'efficacia del PNR, che fa riferimento al piano manifattura Italia, all'aggregazione tramite rete d'impresa, al famoso *masterplan*, che dovrebbe essere un punto di forza e di vitalità per il tessuto economico del Mezzogiorno, che, ad oggi, non ha altri strumenti, se non il *masterplan*, per mirare ad una riduzione degli squilibri territoriali. Eppure nell'ultima legge di stabilità era contemplata la possibilità di prorogare per il Sud d'Italia lo sgravio contributivo per i nuovi assunti, possibilità che nel PNR, invece, manca. Secondo quanto annunciato dal ministro Padoan, proprio a maggio, con l'azzeramento della tassa sul *capital gain,* con il sostegno agli investimenti di aziende non quotate e con gli sgravi sugli utili reinvestiti, si dovrebbe avere un enorme slancio (dello 0,2 per cento) Nel DEF, però, si menzionano poche, pochissime volte le micro, le piccole e le medie imprese. Qualcosa si fa per le più innovative e quelle appena nate - le *startup* ma di fatto l'attenzione è rivolta a una minuscola minoranza di questo patrimonio italiano, che il DEF erroneamente continua a chiamare «piccole e medie imprese», escludendo le microimprese anche dalla nomenclatura industriale italiana; un'indifferenza che mette tristezza e che prosegue ormai da anni. Renzi - come fecero sia Monti che Letta - si ostina a non presentare, come è invece suo obbligo, il disegno di legge per le piccole imprese. Eppure tanto potrebbe essere fatto per le piccole, che subiscono pesantemente i danni del contesto normativo, teatro di un imbarazzante favoritismo verso le grandi imprese. Purtroppo da sempre il Ministero dello sviluppo economico è totalmente prono alle grandi imprese come le recenti cronache giudiziarie hanno chiaramente evidenziato, non è da meno; anzi, con Trivellopoli sembra proprio in *pole position*. Anche Renzi è di fatto obnubilato dagli interessi delle grandi imprese e dai freddi dettami europei: tanto quanto i due Governi precedenti o forse di più, a lui, che a tutt'oggi è il Ministro *ad interim* dello sviluppo economico, va addebitato il disfacimento della base imprenditoriale italiana, che quotidianamente è ormai sotto gli occhi di tutti noi. *(Applausi Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, per capire l'affidabilità del livello previsionale del Documento al nostro esame, ho messo a confronto i DEF predisposti dal Governo Renzi durante gli anni del suo mandato. L'analisi dei principali indicatori segnalati (indebitamento netto, debito pubblico lordo e PIL nominale) sono disattesi rispetto alle previsioni formulate nel primo DEF presentato nell'aprile 2014. L'indebitamento netto, che avrebbe dovuto toccare il valore zero tra il 2017 e il 2018 secondo quanto indicato da quel Documento, toccherebbe tale livello verso la fine del 2019, cioè due anni e mezzo dopo, proprio valutando la proposta contenuta nel Documento al nostro esame. Per quanto riguarda il rapporto debito-PIL, il traguardo considerato di sicurezza del 120 per cento fissato dal DEF 2014 per il 2018, ora, slitta al 2019 e registra 3,8 punti in più rispetto a tale previsione. Entrambi questi indicatori si sono potuti allontanare dalle regole europee del Patto di stabilità e crescita grazie alle clausole di flessibilità richieste e, non sempre facilmente ottenute, alla Commissione europea. Eppure, l'aumento del *deficit* e del debito, sia in valori percentuali che in valori assoluti, non sono stati sufficienti a sostenere la crescita del prodotto interno lordo nominale, creando in più una montagna di maggiore spesa. Rispetto alle attese il PIL segna una minore crescita di 18,4 miliardi nel 2016, di 29,9 miliardi nel 2017 e di 34,4 miliardi nel 2018. Fatte queste premesse, assolutamente oggettive, emergono ulteriori dubbi sulla validità delle politiche che il Governo intende portare avanti nel nuovo quadro programmatico. In confronto al tendenziale, il PIL programmatico scenderà di 2,9 miliardi nel 2017 e tornerà a salire, ma solo di 500 milioni di euro, nel 2018, e di 3,8 miliardi nel 2019. Oltretutto, le stime di crescita del PIL nel 2016 sembrano davvero essere troppo ottimistiche, ove confrontate con una pluralità di previsioni indipendenti e come sottolineato anche da molti durante le audizioni. Di conseguenza, tutte le aspettative riportate sugli altri indicatori legati al PIL (in particolare sul *deficit* e sul debito) sono a forte rischio di inattendibilità. Sicuramente, sia per il 2017 che per il 2018, la deviazione sul *deficit* non rientra nel quadro di rispetto dei parametri del Patto di stabilità e crescita, mentre la regola del debito viene disattesa in tutti e tre gli anni presi in esame. Valutando la realtà espressa dai numeri, l'azione del Governo Renzi (tre manovre per complessivi 76 miliardi, che includono il disegno di legge n. 66 e le due leggi di stabilità) è stata non solo inutile, ma addirittura dannosa per lo sviluppo del Paese. Secondo le stime del modello trimestrale della Banca d'Italia, la crescita del PIL sarebbe stata negativa sino alla fine del 2017, in assenza delle politiche monetarie espansive della Banca centrale europea. Anche il *quantitative easing*, con una iniezione di liquidità adesso giunta a 80 miliardi al mese, ha concorso ad attenuare gli effetti negativi della ridotta crescita dei Paesi emergenti ed ha cercato di indurre una indispensabile ripresa dell'inflazione. Fatto assolutamente importante è che l'azione della Banca centrale europea ha inoltre contribuito a ridurre l'onere sul debito pubblico italiano. I minori interessi pagati sui titoli di Stato hanno regalato all'economia del Paese 10,6 miliardi (rispettivamente 3,2 miliardi nel 2014, 5,9 miliardi nel 2015 e 1,5 miliardi quest'anno). Gli imprenditori italiani che hanno riportato i capitali posseduti all'estero per tramite della *voluntary disclosure*, hanno donato all'azione del Governo 3,6 miliardi; 11 miliardi derivano poi da maggiori tasse a carico dei cittadini; e quasi 43 miliardi di maggiore indebitamento netto sono stati utilizzati per coprire le misure adottate nel triennio 2014-2016. Ecco, in poche righe e in estrema sintesi, i numeri del governo Renzi e l'eredità che lascerà a chi prenderà il suo posto. Tra le misure proposte per il 2017 mancano tagli effettivi alla mastodontica macchina della pubblica amministrazione. La *spending review*, peraltro mai realmente attuata dal Governo in carica, sinora è stata fatta a colpi di mannaia concentrandosi sui servizi forniti ai cittadini da Regioni, Province e Comuni (stiamo parlando di circa 7 miliardi) e solo per una piccola parte con tagli alle spese dello Stato centrale. Va ricordato che molte misure hanno coperture temporanee che potrebbero far scattare tra il 2017 e il 2019 clausole di salvaguardia per complessivi 56 miliardi, con aumenti di accise e IVA. le clausole di salvaguardia vengono programmaticamente disattivate, ma non c'è una chiara indicazione su come avverrà tale disattivazione. A chi pensa di fare una nuova manovra tagliando le *tax expenditures* vorrei solo ricordare che, in realtà, esse sono agevolazioni fiscali. al di fuori di eventuali giochi contabili, dico a me stesso - per ricordarlo a tutti i colleghi - che un taglio alle *tax expenditures* (175 miliardi complessivi) equivale ad un aumento della pressione fiscale. Questa politica di aumento di tasse e dei controlli sta già portando alla chiusura di un numero considerevole di piccole imprese. La *tax compliance* (cioè la fedeltà fiscale) si può pretendere solo nel momento in cui il sistema fiscale sia equo e giusto, altrimenti si rischia di trasformare l'Agenzia delle entrate e le società delegate alla riscossione coatta dei tributi in aguzzini persecutori delle imprese. Nel Paese assistiamo al moltiplicarsi della burocrazia anche in ambiti marginali della nostra economia e tale aumento sta spingendo fuori dal sistema produttivo tante realtà imprenditoriali. Considerato che il maggiore recupero tra il 2014 e il 2015, attraverso la riscossione coattiva, genera un risultato positivo di appena 250 milioni di euro, è evidente che il vero problema di questo Paese non è l'evasione ma la burocrazia e il suo costo. Anche su questo tema, però, il Governo non ha alcuna strategia. A chi dice che non ci sono più margini per tagliare le spese dello Stato, voglio ricordare che le mancate semplificazioni della pubblica amministrazione hanno un costo sul nostro sistema produttivo di più di 30 miliardi ogni anno. Con uno Stato più leggero, ogni euro di oneri tolto alle imprese italiane può essere reinvestito dalle stesse in ricerca, sviluppo, strumenti e ammodernamenti tecnologici; in breve in attività economiche, in sostanza in posti di lavoro. Il numero di dipendenti pubblici è pari a 3,2 milioni di unità (un lavoratore su sette in Italia), per un costo di oltre 160 miliardi annui. I casi di assenteismo al Comune di Sanremo, in un museo di Roma, alla questura di Rimini, alla prefettura di Pistoia, alla ASL di Avellino, all'ospedale di Salerno hanno segnalato che ci sono dipendenti da sanzionare disciplinarmente o penalmente (questa è una ma hanno soprattutto evidenziato che esistono piante organiche composte da numeri pletorici, destinate ad alimentare burocrazia inutile. La spesa per i consumi intermedi è di 132 miliardi. Siccome stiamo valutando un Documento di programmazione, si possono prevedere misure che, senza indurre un impatto negativo sul PIL, prevedano una graduale riduzione delle aree grigie della spesa. Vorrei riservare un' ultima piccola riflessione al *jobs act*. Il ministro Padoan ci ha rivelato che il suo omologo cinese ha lodato il nostro *jobs act*, ma vorrei ricordare al nostro Ministro che il tasso di disoccupazione cinese è al 4 le occasioni per creare nuovi posti di lavoro non vengono dalla riforma del mercato: le imprese assumono se hanno prospettive di crescita reali, non se giungono benefici fiscali momentanei o parziali per fare assunzioni. Concludendo, nel DEF in discussione ci viene prospettata la solita politica economica contraddittoria ed incerta del Governo, che si abbandona in accademiche valutazioni macroeconomiche sulla prociclicità o anticiclicità dei provvedimenti da prendere e che continua ancora a perdersi in valutazioni se quelle da adottare siano misure espansive o restrittive. IL DEF che avremmo voluto leggere e che si aspettavano anche i nostri cittadini avrebbe dovuto proporre soluzioni basandosi non sulle consuete previsioni ottimistiche del Governo, ma su proposte realistiche, concrete e responsabili che potessero finalmente affrontare e risolvere i veri problemi del nostro Paese. Signor Presidente, senatrici e senatori, molti aspetti del DEF sono già stati affrontati dai miei colleghi, ma vorrei ancora sottolineare tre temi, il primo dei quali riguarda la neutralizzazione della clausola di salvaguardia, di cui molti hanno parlato, ed in merito alla quale desidero Il DEF 2016 prosegue la strategia di programmazione economica degli anni scorsi, il cui obiettivo è il rilancio della crescita e dell'occupazione. Dopo tre anni consecutivi di contrazione, l'economia italiana è tornata a crescere nel 2015, ma i segnali di ripresa sono ancora deboli e incerti, anche per il quadro internazionale economico. Quindi fa bene il Governo a proporre di sterilizzare le clausole di salvaguardia, che diventerebbero operative nel 2017 e che rappresenterebbero lo 0,9 per cento del PIL: è una proposta coraggiosa che assorbe una grande quantità di risorse della manovra ma va nella direzione giusta e prosegue la programmazione impostata già nel 2015. È una manovra, per così dire, a basso impatto comunicativo sulla popolazione, che non ne coglie un effetto diretto, perché si tratta di non applicare una misura di tassazione in ma sappiamo che avrebbe effetti sicuramente negativi sulla ripresa della domanda interna. In ogni caso, è anche una buona risposta a chi l'anno scorso pensava che, dopo aver sterilizzato le clausole di salvaguardia per il 2016, non saremmo riusciti a farlo negli anni a seguire. Anche la copertura che avevamo individuato l'anno scorso era stata criticata, ma ce l'abbiamo fatta e ce la faremo anche quest'anno. Veniamo al secondo punto: la capacità previsionale di questo Governo e dei DEF che non ha eguali rispetto a tutti i Governi precedenti di quest'ultimo periodo.

«Rispetto ad un anno fa la ripresa dell'economia italiana si è effettivamente concretizzata e la disoccupazione ha cominciato a ridursi, così che nella media dell'anno la crescita del PIL è risultata sostanzialmente in linea con le previsioni». ancora: «L'Italia nel 2015 è uscita dalla recessione e il PIL è aumentato dello 0,8 com'era stato previsto. La variazione in termini nominali ha superato le aspettative dell'1,5 per cento e l'indebitamento si è collocato

ma anche nel saper prudentemente definirli, tenendo conto di valutazioni, come quelle dell'Ufficio parlamentare di bilancio, organismo di supporto indipendente, che pure quest'anno ha prodotto una relazione che, oltre a essere obbligatoria, è anche estremamente utile. «Il quadro macroeconomico tendenziale appare, per le variabili di crescita e inflazione, sostanzialmente in linea con le previsione del *panel* UPB».

le indicazioni del Governo si allineano in generale in prossimità del limite superiore dell'intervallo previsto dalle stime, ma pur sempre all'interno del *range* individuato. A seguito dell'analisi, l'Ufficio parlamentare di bilancio ha trasmesso il 1° aprile la propria lettera di validazione delle previsioni macroeconomiche tendenziali per gli anni 2016-2019. In più, il 18 aprile ha validato anche il quadro macroeconomico programmatico 2016-2019, pubblicato nel DEF, e ne ha trasmesso l'esito al MEF. Solo un accenno alle autonomie locali: l'ANCI, nelle audizioni sul DEF, ha espresso una valutazione complessivamente positiva sul Documento di economia e finanza. Questo non vuol dire che si sono risolti tutti i problemi con le autonomie - sul tema insisto sempre sulla necessità di una revisione complessiva del sistema di finanziamento delle autonomie locali per ridare loro piena autonomia - ma sicuramente l'ANCI si è espressa in termini favorevoli. Concludo, signor Presidente, con la convinzione che anche il DEF 2016, orientato al rilancio della crescita e dell'occupazione, centrerà i suoi obiettivi. Dipenderà dalla capacità del Governo, ma anche da quella di tutti noi nel garantire il dettaglio di queste linee nella legge di stabilità del 2017.

proposta di risoluzione n. 100, presentata dai senatori Zanda, Schifani e Zeller. Sono inoltre pervenute alla Presidenza, sul Documento di economia e finanza 2016, le proposte di risoluzione

un segnale di grave pericolo di disastro ambientale, di proporzioni decisamente rilevanti. Stiamo parlando di inquinamento di acqua potabile.

dall'Unione europea, ed è posto in una località che si chiama Oliero, vicino ad Asiago, in provincia di Vicenza. Qual è il pericolo? Qualcuno è stato sufficientemente avveduto - non voglio usare altri aggettivi - da autorizzare prima, costruire poi e portare a compimento una grande discarica, che si chiama Melagon, che contiene rifiuti di tutti i tipi,

di una montagna carsica, che è un gruviera e che naturalmente è sottoposta a un processo di erosione e consumazione. È una montagna che naturalmente

arriveremo a un punto in cui il tetto, sopra il quale è posta questa discarica, crollerà e i rifiuti precipiteranno all'interno della montagna e arriveranno a questo bacino, che è il secondo più grande d'Europa e che può dare 300 litri di acqua al giorno per quattro milioni di italiani. Ripeto: abbiamo una discarica enorme posta sopra un monte che è un gruviera e che

che hanno bisogno di bonifica se vogliamo evitare domani una catastrofe annunciata. Non diciamo poi che non lo sapevamo.